"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, è un grande onore e una grande emozione per me ricordare oggi Luciano Guerzoni, a Modena "il senatore" per antonomasia. Luciano Guerzoni, che era nato a Modena nel 1935, ci ha lasciati il 10 agosto scorso. La sua vita è stata caratterizzata da un costante impegno,

Nei ricordi dei tanti che, molto più di me, hanno avuto l'opportunità di frequentarlo, emerge con forza, come fatto distintivo della sua persona, la capacità di coniugare la volontà di coltivare la memoria, perché è dalla memoria che nasce la consapevolezza anche del presente, l'attenzione al quotidiano, che va interpretato e in cui bisogna costantemente operare, e il progetto per il futuro, che è il traguardo dei nostri valori e della nostra identità. Da questi ricordi emergono anche due tratti costanti alla base della sua azione: la militanza antifascista, fondata sulla acuta consapevolezza che quello che è accaduto potrebbe nuovamente accadere, e l'attenzione ai giovani, alle loro aspirazioni, ai loro diritti, in altre parole, al loro futuro. È impossibile dare conto dell'intera opera di Luciano Guerzoni. Mi limiterò a ricordare alcuni elementi essenziali della sua azione in quattro campi principali: nazionale partigiani d'Italia (ANPI). Nel partito Luciano Guerzoni ha operato come militante: una militanza di servizio per la sua costante disponibilità all'ascolto e al confronto e, al tempo stesso, una militanza di responsabilità, per i diversi ruoli direttivi che è stato chiamato a svolgere, sia a livello locale (è stato anche segretario cittadino del PCI di Modena) che a livello nazionale. Fra le costanti della sua azione politica dentro al partito ricordo la volontà di conoscere e approfondire e l'impegno nella formazione dei giovani, a partire da quando era giovane lui stesso. Come amministratore Luciano Guerzoni è stato consigliere, comunale prima e regionale poi, e alla guida della Regione Emilia-Romagna fra il 1987 e il 1990. Sono anni in cui ha agito come protagonista del riformismo emiliano e del buon governo dei nostri territori. È stata sempre forte in lui la cultura delle autonomie locali e dello stretto legame che deve esistere fra amministrati e amministratori. È lui stesso a ricordare come particolarmente significative di questo periodo due leggi di grande rilevanza sociale e culturale. L'una è relativa alle scuole dell'infanzia, che ha allargato e qualificato il servizio e contribuito ad affermare il particolare modello integrato pubblico-privato che ha garantito una presenza capillare del servizio sul territorio regionale facendo, per citare le sue parole, delle scuole per l'infanzia vere e proprie agenzie educative sul territorio; nell'altra, la legge paesaggistica, si sviluppa una concezione moderna dell'uso del territorio e della tutela delle sue parti più pregiate. In Parlamento Luciano Guerzoni è stato eletto al Senato nel 1992, per essere poi riconfermato fino al 2006. Quattro legislature in cui ha mantenuto un continuo e fruttuoso rapporto con il suo territorio di provenienza per ascoltarne i bisogni e le domande e farsene interprete a livello nazionale. grazie Voglio ricordare, in particolare, sia il suo ruolo di Vice Capogruppo, per il suo Gruppo parlamentare, sia i ruoli che ha ricoperto nelle Commissioni in cui ha messo a frutto le sue conoscenze e la sua esperienza di amministratore, in particolare come Presidente della Commissione sulle questioni regionali e di quella finanze e tesoro. Particolarmente significativo nel suo percorso di coerente antifascista è stato il ruolo svolto come Vice Presidente nella Commissione di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Una Commissione assai importante, che, fra l'altro, condusse all'acquisizione di un materiale documentale di grande importanza relativo alla vicenda nota come "armadio della vergogna", al cui occultamento sembrano aver contribuito, secondo le connessioni riscontrate in sede parlamentare, anche direttive di ordine politico. Un impegno, quello di Guerzoni nella Commissione di inchiesta, in linea con quello che lo ha sempre animato a conoscere e far conoscere, far ricordare, impedire che ci si dimentichi cosa sono stati il fascismo e il nazismo in Italia e in Europa. Nell'ANPI, l'impegno di Luciano Guerzoni diventa prioritario quando viene eletto nel 2006 tra i componenti del comitato nazionale ANPI e poi, dal 2007, entra nella segreteria nazionale. È qui che mette a prova le sue note capacità organizzative, contribuendo fortemente al rilancio operativo dell'intera associazione, non solo con le sue idee, ma anche garantendo la sua presenza fisica su tutti i territori

Voglio citare fra tutti la manifestazione, organizzata assieme anche alla CGIL, del 1° maggio a Portella della Ginestra, nel 2010, in ricordo della strage del 1° maggio 1947 quando, durante una manifestazione contro i latifondisti, furono uccise undici persone dalla banda di Salvatore Giuliano. Anche nell'ANPI prosegue la sua attenzione e, quindi, la sua attività nei confronti dei giovani. Voglio ricordare, ad esempio, quando, in occasione del 150° dell'unità d'Italia, organizzò un raduno giovanile nei luoghi dell'esilio di Garibaldi, presentandolo con queste parole: «L'incontro tra i giovani avrà il valore umano della conoscenza, sarà occasione di un interscambio culturale e politico, consentirà la possibilità di costruzione di fruttuosi rapporti all'interno dell'associazione». Dal 2012 fu chiamato a ricoprire la carica di vice presidente vicario della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e partigiane e non si arresta per niente la sua progettualità. Da ultimo, si è adoperato molto per la informatizzazione di tutti i fascicoli del fondo Ricompart, custodito presso l'Archivio centrale dello Stato, per rendere pienamente fruibile a studenti, docenti e studiosi il materiale del fondo. È un lavoro che l'ANPI, oggi presente con una qualificata delegazione, che saluto, ad assistere a questa commemorazione, intende proseguire con determinazione. Ho conosciuto personalmente Luciano Guerzoni solo nel 2016, in occasione dell'impegno comune per il no al recente *referendum* costituzionale. Ho potuto apprezzarne le doti di persona equilibrata e appassionata al tempo stesso, diretta nei rapporti, capace di mettere a proprio agio l'interlocutore, disponibile al cambiamento ma fortemente radicata nei valori.

convissuto e condiviso l'esperienza del Consiglio comunale a Modena, dal 1975 al 1980, quando in quel Consiglio comunale sedevano ventinove comunisti eletti nel Partito Comunista Italiano e dodici democristiani Nel 1980, insieme siamo andati in Consiglio regionale, con una analoga situazione: ventinove comunisti e dodici democristiani. Guerzoni, sia in Consiglio comunale che in Consiglio regionale, già appariva per quello che è sempre stato nella sua vita: una persona seria, appassionata dell'attività che svolgeva e di poche parole ma, come nella tradizione dei suoi grandi colleghi che ho conosciuto, quando una parola la dava, la manteneva. Ricordo, in Regione Emilia-Romagna, due altri grandi protagonisti di quella grande stagione, Decimo Triossi e Giorgio Ceredi, uno di Ravenna e l'altro di Forlì, forse qualcuno di voi ha conosciuto. Giorgio Ceredi, grande assessore all'agricoltura, diceva: hai ragione, te la posso dare; oppure: ritengo che tu abbia torto; la terza ipotesi era: hai ragione, ma per ragioni politiche non te la posso dare. con grande trasparenza, con grande chiarezza e con grande autorevolezza. Decimo Triossi ricordava come l'impegno di funzionario del partito fosse allora assunto con spirito di sacrificio, di rinuncia e nella prospettiva (con una battuta che allora andava di moda) di persone che dividevano il mondo in due categorie: chi era comunista e chi lo sarebbe diventato. Vi era sempre, quindi, questa

incarico che mantenne con l'usuale serietà, con la disponibilità, però, a parlare con tutti e con un approccio rigoroso e religioso di rispetto delle istituzioni.

irrevocabilmente e ci subentrarono altri colleghi, in attesa che vi fossero le elezioni. Soltanto dopo scoprimmo (e ne ridemmo, un po' amaramente) che in quasi tutte le Regioni di Italia i nostri colleghi avevano fatto finta di dimettersi e quindi, se eletti, erano entrati in Parlamento, se non eletti, avevano perso in qualche cassetto le dimissioni che avevano prestamente ritirato. Vi assicuro, però, che in Emilia-Romagna a nessuno, maggioranza o opposizione, democristiano o comunista, era passato neanche per l'anticamera del cervello di non rispettare scrupolosamente le regole dettate per le elezioni. poi ci siamo un po' persi di vista, nel senso che, per il gioco della politica, come io ero minoranza quando lui era maggioranza in Consiglio comunale e, quando eravamo in Consiglio regionale, lui era Presidente mentre io ero all'opposizione, così a Roma ci siamo

La vocazione che aveva per la politica attiva l'ha trasferita nell'ANPI, perché ci credeva, perché fino all'ultimo ha servito la causa in cui credeva. E allora, come ho detto anche a Modena, quando molti liquidano con superficialità la Prima Repubblica e gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta dico: magari ci fossero nella Seconda e nella Terza Repubblica uomini come Luciano Guerzoni, che onorano la parte politica che hanno servito e di cui hanno fatto parte! *(Applausi).* Signor Presidente, cari colleghi, cari familiari e amici dell'ANPI presenti in tribuna, non nascondo, come la collega Guerra, sia l'orgoglio che l'emozione di parlare in quest'Aula, dove Luciano ha operato per tanti anni. A Modena Luciano Guerzoni era per tutti "il senatore"; non importa se non ricopriva più quella carica da qualche anno o chi altri in quel momento fosse a Palazzo Madama. Luciano Guerzoni era "il senatore", perché quell'appellativo se l'era guadagnato sul campo, per la sua autorevolezza, per la sua serietà, per la sua passione, per la sua competenza e anche per il suo impegno indefesso. Chi voleva parlargli, per qualsiasi ragione o qualsiasi fosse la sua idea politica, non aveva che da chiedere un appuntamento. Lui in ufficio, nella federazione del PCI di Modena, passava tutte le settimane, sempre, e ne faceva un punto d'onore di trovare il tempo per ascoltare tutti. Il mio conterraneo, senatore per tre legislature, ma anche Presidente della Regione e vice presidente nazionale dell'ANPI, ci ha lasciato, com'è stato detto, il 10 agosto scorso. Per me, giovane amministratore, è stato un esempio; da parlamentare, un modello. La sua passione per la politica lo ha guidato fin da giovanissimo, quando, già iscritto al Partito Comunista, per pagarsi gli studi universitari aveva lavorato come operaio alla Fiat e alla Maserati, dove divenne programmatore Ben presto cominciò a ricoprire incarichi sempre più di responsabilità all'interno del partito modenese: divenne consigliere comunale a Modena, poi consigliere regionale, poi, come si è detto, apprezzato Presidente della Regione, espressione di quel riformismo emiliano che tanto ha dato al nostro Paese. Nel 1992 si candidò al Senato, con il Partito Democratico della Sinistra; dopo essere stato eletto, divenne Vice Capogruppo del PDS. Le ultime due legislature le svolse nelle file dei Democratici di Sinistra. Da lui, tutti quelli come me, cresciuti a Modena nella FGCI degli anni Ottanta e Novanta e appassionati della politica, hanno imparato cosa fosse il legame con il territorio per un parlamentare: l'essere sempre a disposizione, il rapporto sano con gli interessi che si dovevano rappresentare, anche al di là delle appartenenze e degli steccati politici, per il bene di quella comunità, nel rapporto con tutte le sue rappresentanze. Imparammo anche tanto altro dalle sue azioni e dalle sue parole, perché non si sottraeva mai al confronto e all'incontro, soprattutto con noi giovani. Nel tempo era diventato anche un amico e - se posso permettermi di sottolinearlo - la stima era diventata reciproca. Assieme al senatore Giuliano Barbolini fece la scelta, allora non certo facile, anche di sostenermi nella sfida per la segreteria provinciale dei Democratici di Sinistra modenesi nel congresso del 2001. La frequentazione è continuata negli anni e il suo senso della politica come servizio per il bene comune, del modo giusto con cui le cose devono essere affrontate, non è mai cambiato, neppure quando non rivestiva più incarichi di partito. A inizio di questa legislatura, nel nuovo ruolo di vice presidente dell'ANPI, cercò di trasmettere a me e ad altri senatori del Partito Democratico il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze parlamentari sul tema della memoria del Novecento, a partire dai risultati che ottenne con il cosiddetto "armadio della vergogna", che riuscì, assieme ad altri, ad acquisire e ad aprire, scoprendo gli atti e i documenti sulle stragi naziste compiute nel nostro Paese durante il Secondo conflitto mondiale. Anche quando le posizioni politiche divergevano, com'è stato sul *referendum* del 4 dicembre scorso, non è mai mancato il confronto schietto e sincero. Ricordo che proprio l'anno scorso, in occasione della festa provinciale

Mi disse: «Chiedi prima ad Alfonsina Rinaldi, Stefano. Sai, lei era segretario della federazione del PCI in quegli anni. Poi, se non può, vengo io. Sai, sono un po' stanco, ma vengo volentieri». È vero, era un po' stanco negli ultimi tempi, a causa anche della malattia, ma sempre attentissimo a tutto quanto stava accadendo, all'evolversi della situazione locale come di quella nazionale. Il senatore Luciano Guerzoni è stato davvero un punto di riferimento per tante generazioni di una comunità politica che è cambiata molto (certo, e non poteva essere altrimenti) in questi anni. Ci mancheranno tanto i suoi consigli e le sue riflessioni, ma anche i suoi incoraggiamenti e il suo sostegno, e nelle prossime settimane quella comunità, a partire dall'ANPI, so che gli tributerà l'omaggio che gli spetta. In conclusione, a nome del Gruppo del Partito Democratico, voglio esprimere la vicinanza e le sentite e commosse condoglianze ai familiari qui presenti e dire: ciao Luciano, grazie per tutto quanto ci hai dato e lasciato.

Anche personalmente ricordo l'impegno, la solidità e la concretezza del senatore Guerzoni che in tante occasioni ho incontrato nelle Aule parlamentari. In sua memoria invito l'Assemblea

di digerire un momento di commozione comune e di ricordo di un collega. È un po' come nel mondo dello spettacolo: lo spettacolo deve andare avanti. Mi scuso quindi se stavo parlando con il collega, continuando privatamente il ricordo comune di un grande personaggio.

Facciamo un gioco: se tu fossi stato al Governo, cosa avresti fatto? Probabilmente, se fossi stato al Governo, nel momento in cui veniva presentato l'emendamento riguardante i cani e i cavalli, mi sarei rimesso avrei interpretato la stragrande maggioranza del Senato - io la penso così - che aveva trovato una concordia sull'eliminazione,

È chiaro che questa loro specializzazione è il frutto del lavoro degli istruttori e di un esercizio continuo che insegna loro a lavorare o che insegna ad altri animali a svolgere attività, come quelle olimpioniche che sicuramente, nella civilissima Inghilterra, vengono svolte anche a scopo

operando in maniera tale che venga garantito il benessere animale, facendo più controlli - ci mancherebbe altro, più controlli ci sono e meglio è - ma anche governando la questione senza mettere a rischio il lavoro di 6.000 persone e senza - lo ripeto per l'ennesima volta ed è una delle ragioni della nostra astensione - che un Parlamento possa cancellare Fellini, possa cancellare il grande Totò,

donne. Un Parlamento non può fare questo, perché vorrebbe dire non fare un passo in avanti, ma regredire rispetto ad intere generazioni di persone che si sono appassionate e ancora oggi sono appassionate,

l'esaltazione, sempre fatta dalla dottrina della Chiesa, del fatto che non ci debba essere contrapposizione fra uomini e animali ma un rapporto di collaborazione. Queste sono le ragioni per le quali noi daremo un voto di astensione

la qualità degli interventi e la passione che molti colleghi hanno messo in discussione generale sono la riprova di quanto siano sentiti il tema e il provvedimento. Certo, resta il rammarico di una legge delega che giunge all'ultima curva della legislatura. Forse si poteva fare prima, per portare così a compimento il buon lavoro di questi anni, con il quale si è dato un impulso significativo all'intero settore culturale e artistico e che, come ha ribadito più volte il Ministro, deve puntare a essere una delle voci più rilevanti dell'economia del nostro Paese. In questo quadro, restiamo dell'avviso che dobbiamo rafforzare gli strumenti e le risorse anche a favore del volontariato culturale, non solo per le implicazioni di crescita economica, ma anche perché l'impegno del volontariato culturale forma e consolida la coesione di una comunità viva e responsabile, che partecipa e valorizza le relazioni, che favorisce l'integrazione e l'inclusione sociale, anche nei luoghi più piccoli o periferici. In discussione generale ho già illustrato quelli che, a nostro avviso, sono i punti di forza e gli elementi di criticità della legge. In questa sede, non mi resta che rinnovare l'invito al Governo a farsene carico con la prossima legge di bilancio. In Commissione cultura, anche attraverso gli ordini del giorno che ho sottoscritto e promosso, il Governo ha ribadito un impegno concreto che mi auguro rispetterà; l'ha chiesto con convinzione anche la relatrice Di Giorgi, che ringrazio. Anzitutto dobbiamo rendere permanente la possibilità per i contribuenti di scegliere le associazioni culturali a cui assegnare il due per mille nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di una possibilità di finanziamento a cui le associazioni e l'intero mondo del volontariato guardano con favore, anche perché le sollecita a lavorare sempre più e meglio, in un rapporto di ancora maggiore sinergia con i cittadini e con il territorio. Ma occorre anche introdurre agevolazioni fiscali per le realtà bandistiche, corali, filodrammatiche, coreutiche e folkloristiche per l'organizzazione di corsi di formazione, per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici che effettuano prestazioni a carattere intermittente. E si deve pensare a una qualche forma di detrazione a favore delle famiglie per l'iscrizione dei figli a corsi di formazione, alla stessa stregua di quanto accade per lo sport. Vi è, infine, la necessità di una revisione della disciplina del diritto d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal vivo di brani musicali. A riguardo ho presentato uno specifico ordine del giorno, e ringrazio il Governo e la relatrice per averlo accolto, così come sono stati accolti quelli analoghi presentati dai colleghi. Può sembrare una piccola lista della spesa, ma non lo è. Chi, come me, conosce da sempre il mondo del volontariato culturale sa bene quanta passione, impegno e competenze vengono messi in campo ogni giorno, e di questo dobbiamo essere grati a tutti coloro che continuano a spendere gratuitamente le loro energie. E so quante siano le difficoltà nel portare avanti attività così meritorie, che hanno una lunga tradizione nel nostro Paese e che sono fondamentali sia per la qualità della vita delle nostre comunità, che per la promozione turistica, che per l'immagine dell'Italia nel mondo. Per questo l'invito che rivolgo all'intero Governo è di rafforzare questi ambiti, soprattutto sul terreno delle risorse loro destinate. Non ricevono più nulla dal FUS e ben poco dagli enti locali; vivono spesso solo della buona volontà dei loro sostenitori e adesso attendono che alle buone intenzioni seguano i fatti. Accanto al mondo del volontariato bisogna poi mettere al centro i talenti. C'è una generazione creativa e innovativa che è depositaria di nuovi saperi e conoscenze, che ha competenze importanti, in grado di produrre anche valore economico e occasioni di lavoro qualificato. Proprio ieri alla Camera è iniziata la discussione su un provvedimento per le imprese culturali e creative, le *start up* giovanili, con cui si prevedono sgravi dal punto di vista tributario e degli ammortamenti. È una proposta interessante e speriamo davvero possa concludere il suo *iter* prima della fine della legislatura. In conclusione, il nostro auspicio è che questa delega, che affronta davvero tante questioni, che mette ordine e dà una più solida cornice normativa a tanti settori che la attendevano da tempo, sia un ulteriore tassello perché la cultura sia sempre più centrale anche per le ricadute economiche e per aumentare la competitività del nostro Paese. Ma per farlo dobbiamo tenere conto della cultura in tutte le sue espressioni, da quelle più alte a quelle più popolari, da quelle della tradizione a quelle che producono nuovi saperi, creatività e innovazione. Tutte devono essere messe nella condizione di esprimere il loro potenziale, contribuendo così a rafforzare i dati positivi sulla crescita del Paese. È con questo auspicio, ringraziando ancora la relatrice e i colleghi della Commissione cultura, che dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento. Signor Presidente, il provvedimento in esame interviene in un ambito fondamentale per ogni Paese, avendo quale oggetto il settore della cultura, un mondo in cui l'Italia è storicamente all'avanguardia con le proprie produzioni. Investire in cultura non può che rappresentare motivo di orgoglio, specialmente se ciò avviene in un difficile contesto economico-finanziario, ed è per questo motivo che dispiace particolarmente trovarsi dinanzi all'ennesima occasione sprecata. Le misure previste da questa legge delega sembrano più mirate a garantire la mera sopravvivenza del settore che non a puntare su un vero e proprio rilancio del mondo dello spettacolo italiano, universalmente noto e ammirato. L'intento dì realizzare una disciplina organica dello spettacolo è certamente encomiabile, ma in realtà il provvedimento in esame appare eccessivamente vago nel delineare ambiti e modalità su cui il Governo dovrà cimentarsi con i decreti delegati. Non si può non ricordare che parliamo di un argomento che è per noi innanzitutto storia e tradizione e dovrebbe quindi essere concretamente e adeguatamente valorizzato. La tradizione, infatti, resta tale se viene continuamente rivitalizzata; se non è incentivata, diventa una leggenda, solamente un ricordo. E questo provvedimento pecca soprattutto per aver mancato la possibilità di fare dello spettacolo e delle varie forme d'arte che esso comprende un settore su cui soprattutto i più giovani potessero investire per il proprio futuro, cosa che invece è stata in parte prevista con la recente approvazione della legge sul cinema e l'audiovisivo, di cui il testo oggi in esame è uno stralcio. Quello dello spettacolo è un settore in crisi che bisogna risollevare con sovvenzioni e incentivi mirati e diretti a sostegno delle attività artistiche, con una programmazione sistemica delle misure e delle modalità in grado di avere effetti concreti nel lungo periodo. Qui si prevede, invece, un'ulteriore complicazione burocratica per l'accesso ai fondi con la sostituzione della vecchia consulta per lo spettacolo con il consiglio superiore dello spettacolo, cui si affida, tra le altre cose, anche il compito

e vaghezza circa gli interventi a favore delle accademie, il cui ruolo è invece storicamente di cruciale importanza per questo settore. Le accademie italiane hanno infatti sempre rappresentato un'avanguardia, anche nel più ampio contesto internazionale, e avrebbero dunque meritato una maggiore attenzione per rilanciarne le attività. Anche i circhi non hanno trovato la giusta e meritata attenzione in un provvedimento che sembra non tenere minimamente in considerazione un'importante e antica tradizione che, al pari delle altre forme d'arte, richiede impegno e dedizione, oltre che particolari capacità non solo fisiche, sviluppate in scuole e istituti per la formazione nelle singole discipline. Quello dei circhi è, infatti, un universo artistico tra i più ampi, che racchiude dagli attori maestri di comicità agli atleti, dai ginnasti agli illusionisti: insomma una parte decisamente consistente di quello che viene comunemente definito come mondo dello spettacolo. Le misure adottate per il mondo circense sembrano, invece, destinate esclusivamente a comprometterne l'attività e non vi sono iniziative meritevoli di nota per sostenerne e incentivarne la diffusione. Si è voluto associare i circhi solamente al controverso utilizzo degli animali in determinati spettacoli, ponendosi l'obiettivo di inasprire le normative attualmente in vigore, che sono forse già eccessivamente stringenti. Tutto il resto degli spettacoli che si svolgono sotto i celebri tendoni è stato letteralmente ignorato e nulla è stato previsto per la loro valorizzazione. La stessa idea di rilanciare lo spettacolo italiano anche all'estero non sembra fare adeguatamente i conti con il contesto multiculturale che si delinea in maniera sempre più marcata nelle società moderne e che dovrebbe essere inteso anche come momento di comune arricchimento, In conclusione, il testo oggi in esame appare carente nella stessa previsione di rilanciare un comparto che, se adeguatamente incentivato, darebbe un ritorno importantissimo sia in termini economici che culturali.

Presidente, quello oggi alla nostra attenzione è un provvedimento di delega, attraverso il quale il Parlamento indica al Governo i principi cui dovrà attenersi nella ridefinizione delle norme che riguardano un settore fondamentale per lo sviluppo culturale e il mantenimento delle tradizioni del nostro Paese, che è il settore dello spettacolo dal vivo. Nel testo rinveniamo princìpi condivisibili, tratti dalla necessità di aggiornare, regolare, rivedere, svecchiare e innovare un settore multiforme e ricco di creatività.

sicura ragionevolezza, onde pervenire a un provvedimento quanto più condiviso. Tra l'altro, la mole di audizioni

Ho ascoltato con attenzione gli interventi che si sono susseguiti durante la discussione generale e ho potuto giudicare taluni di essi importanti, chiarificatori e pertinenti. Nei pochi minuti a mia disposizione vorrei, però, poggiare l'accento su un aspetto che reputo fondamentale in tema di

più estremista e i circensi, riguardo l'utilizzo degli animali nei circhi. Accolgo con favore le istanze dei circhi e del loro personale, che legittimamente sostengono che senza animali un circo non può sopravvivere. Alcune famiglie circensi hanno provato a metter su spettacoli completamente privi di animali, ma hanno toccato con mano quasi l'azzeramento dell'*appeal* dei loro spettacoli. *Ergo*, non basterebbero solamente acrobati, *clown* e giocolieri, ma la tradizione popolare più autentica del circo rende indispensabile la presenza degli animali. Il pensiero, tuttavia, non va solamente ai lavoratori del circo che in siffatta maniera rischiano la disoccupazione. Il mio ragionamento va oltre e investe l'essenza stessa dello spettacolo circense. Dovremmo scomodare la nutrita filmografia sulla magia del circo per rammentare a noi stessi il messaggio di grande umanità che ci perviene dalla variopinta tenda del circo, con tutta la semiologia dell'abbandono, della solitudine, dell'alternanza degli stati d'animo tra allegria e tristezza. il tema non è la presenza o meno degli animali nel circo. La questione riguarda semmai il loro trattamento. Personalmente ritengo che qualunque addestratore abbia necessità di entrare in empatia con l'animale e non abbia alcun interesse - a meno che non si tratti di un bruto ignorante - a trattar male l'animale che si esibisce nei suoi numeri. E allora è lì che bisogna intervenire, ossia sui controlli e sul rispetto delle norme e dei protocolli già esistenti sul punto. Vogliamo inasprire le sanzioni in caso di violazione? Bene, facciamolo. Vogliamo implementare i controlli sui circhi in ogni piazza? Benissimo. Vogliamo puntare su un innovativo protocollo d'intesa fra ASL, enti di protezione e istituzioni per l'utilizzo degli animali nello spettacolo e nello sport che, nel rispetto della normativa vigente, responsabilizzi ulteriormente gli operatori? Non chiediamo di meglio. Non mi si venga però a dire che non è etico impiegare gli animali nel circo, perché, se così fosse, allora dovremmo bandire l'ippica, il *dressage*, l'addestramento dei cani per ciechi, l'addestramento dei cani per il salvataggio in acqua o tra le macerie di un terremoto o di una slavina. Anche questi animali vengono addestrati e fatti lavorare per lo più in posti disagiati e ricchi di insidie. E che dire degli animali impiegati per le produzioni cinematografiche? A quelli è consentito essere addestrati per lo scopo? Mi pare ci muoviamo in un campo minato da manifesta disparità. Mi sembra quindi che i sostenitori più accesi dell'eliminazione degli animali nei circhi siano anche quelli che forse sanno meno di etologia e addirittura meno conoscono le caratteristiche comportamentali degli animali che nascono in cattività. Ebbene, non posso non rammentare a quest'Assemblea il carico di ilarità e spesso di ironia, la sufficienza che hanno destato le prese di posizione del senatore Giovanardi, che ha sostenuto ragioni di buon senso e la necessità, in buona sostanza, di prestare attenzione e aprire le orecchie a quanto la scienza, richiamata anche dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, ci induce a considerare riguardo, appunto, il comportamento degli animali. Pare che questa Assemblea non abbia voluto

Ci si dimentica di una cosa non indifferente, e cioè che in un mondo così tecnologizzato, urbanizzato, che ha superato la civiltà contadina, che oggi si direbbe postindustriale, il contatto con circhi e zoo (oggi chiamati bioparchi) diventa l'unica possibilità per buona parte della popolazione (specialmente delle fasce giovanili e infantili) di poter vedere dal vivo animali che solo in televisione o nell'immaginazione possono conoscere. E la cosa non mi appare indifferente, tanto più che la globalizzazione, con effetti di mercificazione e omologazione verso il basso, sta colpendo oggi pesantemente anche i settori della cultura, determinando la necessità di riscoprire i valori autentici alla base della tradizione, e quindi della cultura popolare e dell'identità di una comunità nazionale. Mi sembra allora un accanimento incomprensibile nei confronti di una piccolissima comunità, quella circense, che forse non è adeguatamente difesa, perché non è produttrice di voti come i gruppi animalisti più estremisti, né questa né questa comunità si presta a operazioni commerciali che oggi prevalgono anche nel grande *business* milionario del cibo per animali. Auspico quindi che sull'argomento la partita non sia chiusa e il Governo utilizzi un discernimento equilibrato sulle prospettive che tenga conto dell'afflato che tenga conto dell'afflato levatosi in quest'Aula a favore delle attività circensi animate dagli animali, in particolare dai cani e dai cavalli. Per il resto, il provvedimento

Ma - come sempre accade per le leggi delega - dovremo attendere i decreti di attuazione per giudicare l'impatto concreto del provvedimento. Siamo pertanto compiaciuti del contributo offerto dalla mia parte parte politica e dalla mia presenza in Commissione sui riconoscimenti che finalmente giungeranno al variegato mondo delle tradizioni popolari,

culturale, rappresentato dal compito fondativo di divulgare i repertori musicali in giro per la Penisola, su e giù per città, paesi e contrade, a beneficio delle popolazioni residenti, che mai avrebbero e tuttora non hanno l'occasione di assistere a grandi esecuzioni lirico-sinfoniche. La delega al Governo comprende anche le rappresentazioni storiche e i cortei storici, la danza, il jazz, la musica giovanile, la prosa e il dramma. Apprezziamo anche i contenuti della delega sull'estensione dell'Art bonus al settore dello spettacolo. Avremmo voluto, Presidente - mi avvio davvero alla conclusione - che l'Art bonus fosse

questo tipo di editoria. Per queste ragioni, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo delle Grandi Autonomie e Libertà, il nostro voto sarà di astensione. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, come Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, sin dall'esame in 7a Commissione di questo provvedimento, ci siamo accostati ad esso con spirito propositivo, nell'obiettivo di migliorare un impianto che abbiamo giudicato nel complesso soddisfacente. In coerenza con questo atteggiamento, abbiamo presentato alcune proposte emendative che sono state accolte e hanno riguardato, *in primis*, la tutela dei lavoratori impiegati nel mondo dello spettacolo, con particolare riferimento agli aspetti retributivi; poi l'insieme di condizioni atte a favorire la diffusione di opere di giovani artisti e compositori emergenti, e infine la più ampia fruizione dei contenuti dello spettacolo dal vivo da parte delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia, in linea con quanto previsto anche dalla legge sul cinema e l'audiovisivo. Una attenta valutazione delle domande e delle aspettative che vengono dal mondo dello spettacolo - domande che una nuova forza politica, sensibile al mondo del lavoro e alla tutela e allo sviluppo della cultura, quale noi siamo, ha il dovere di raccogliere e di rappresentare - e un confronto approfondito con i sindacati di categoria, in particolare con la segreteria nazionale della CGIL-SLC, settore produzione culturale, ci hanno spinto a sottoscrivere e sostenere otto emendamenti presentati dai senatori Bocchino e Petraglia di Sinistra Italiana, relativi alla situazione e ai problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche, che esprimono un orientamento diverso rispetto a quello del Governo che, appunto, ci siamo sentiti di condividere. Stiamo infatti parlando di un'arte, quella lirico-sinfonica, che illustra, forte di una plurisecolare tradizione, il buon nome dell'Italia nel mondo intero e di un comparto professionale che dà lavoro non soltanto agli artisti, ma anche a migliaia di maestranze necessarie ad allestire gli spettacoli. Com'è noto, una grave crisi ha investito la maggiore parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, che hanno raggiunto un debito complessivo superiore a 300 milioni di euro nel 2012, tanto che nel 2013 è stata disposta la possibilità per le fondazioni di ristrutturare, a certe condizioni, il proprio debito, grazie a un prestito trentennale. Nel corso degli anni, si sono battute le solite vie neoliberiste per cercare di risolvere la crisi debitoria, a cominciare dalla riduzione dei salari dei lavoratori legati alla trattativa di secondo livello, fino ad arrivare all'azzeramento dei corpi di ballo di diverse fondazioni. La riduzione di personale è avvenuta, oltre che per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, mediante incentivi e aperture delle procedure di esubero, anche grazie alla continua e crescente esternalizzazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro. Si è inoltre attuata, mediante una contrazione degli organici a tempo determinato delle orchestre, un'arbitraria rivisitazione di quanto richiesto dalle partiture dei compositori, laddove gli organici stabili non permettevano l'esecuzione di certi repertori. Insomma, per risparmiare si è arrivati a riscrivere addirittura la storia della musica. Nonostante tutti gli sforzi e i sacrifici richiesti e compiuti dai lavoratori - anzitutto dai lavoratori - si è registrata un'ulteriore crescita del debito. Rimane, dunque, una preoccupante situazione di criticità con cinque teatri che hanno il dato patrimoniale negativo, mentre per i restanti tre - su un totale di 14 - il debito è comunque di molto superiore al patrimonio disponibile. Come Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista riteniamo indispensabile aprire una discussione pubblica nel Paese, che parta proprio dal riconoscimento del valore speciale di queste imprese, per poi formulare una proposta atta ad affrontare correttamente le criticità presenti. Sulla scorta di questa impostazione annunciamo il nostro voto positivo al complesso del provvedimento, ma teniamo fermi e abbiamo quindi sostenuto gli emendamenti sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

il dettato costituzionale, che all'articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Non si può promuovere senza lungimiranza e investimenti, capaci di mantenere nel loro prestigio le nostre maggiori istituzioni culturali; di riportare al centro la musica, a partire da quella lirica; ampliando il pubblico e curando la sua competenza; puntando sul territorio, ma al tempo stesso secondo una capacità di intervento di respiro nazionale, così da scongiurare provincialismi e chiusure corporative o di tipo localistico. Ricapitolando - a nostro modo di vedere - bisogna abbandonare una volta per tutte la logica meramente contabile, per non dire mercantile, del pareggio di bilancio; considerare le risorse di un eventuale mecenatismo privato, che deve essere incentivato, come aggiuntive e mai sostitutive dell'impegno pubblico. Bisogna piuttosto procedere con un'oculata e certo sorvegliata politica di investimenti, per rilanciare, nel caso specifico delle fondazioni liriche, al netto dei problemi di controllo delle gestioni, la loro attività. L'obiettivo deve essere la salvaguardia specifica di questi teatri e delle loro capacità artistiche e tecniche, anche tramite la stabilità dei rapporti di lavoro lo ripeto - sono sempre più precarizzati ed esternalizzati. D'altro canto, riteniamo si debba cominciare a ragionare in termini di distretti culturali, così da facilitare l'incontro tra musica colta e fruizione di massa, operando al tempo stesso perché straordinarie competenze tecniche, artigianali

Da qui la portata sistemica della posizione di Articolo 1-Movimento democratico e progressista rispetto al nuovo codice dello spettacolo: appoggio all'insieme della manovra, ma tenendo fermo un punto di vista, che riteniamo indispensabile per implementare la valenza positiva dell'insieme del provvedimento.

Signor Presidente, egregi colleghi, si conclude oggi il lungo percorso del disegno di legge sullo spettacolo dal vivo, inizialmente inserito all'interno del provvedimento sul cinema. Ritengo sia stata una proposta opportuna quella della relatrice, senatrice Di Giorgi, volta all'estrapolazione di questo tema da quel provvedimento: tale proposta, fra l'altro, è stata unanimemente condivisa dalla 7a Commissione All'interno di quel provvedimento, lo spettacolo dal vivo non avrebbe avuto il ruolo e la dignità che ha acquisito con il disegno di legge in esame, come ho già avuto modo di sottolineare nell'intervento in discussione generale. Spesso si parla di leggi non condivise, ma ritengo che questo sicuramente non si possa dire per il disegno di legge n. 2287-*bis*, perché alla decisione che ho ritenuto opportuno citare è seguito un laborioso *iter* in Commissione con numerose audizioni di rappresentanti di tutte le componenti che, a diverso titolo e con diversi ruoli, sono coinvolte nel variegato mondo dello spettacolo; audizioni che hanno consentito di esaminare a 360 gradi tutte le problematiche del settore settore nel quale l'Italia vanta delle eccellenze davvero uniche e universalmente riconosciute. Basti pensare - solo per fare qualche esempio - alla tradizione della lirica italiana o della musica sinfonica o del teatro. Il provvedimento che stiamo per approvare non si limita alle forme maggiormente conosciute in Italia e all'estero, perché dedica grande attenzione ad altre forme che hanno origini meno lontane nel tempo ma che non per questo sono meno valide dal punto di vista della proposta culturale, né meno coinvolgenti dal punto di vista della partecipazione popolare. Mi riferisco al grande sviluppo che hanno avuto negli ultimi decenni le attività artistiche amatoriali come le rievocazioni storiche, i carnevali storici, il teatro, la musica e la danza amatoriali e anche attività non amatoriali ma lavorative come quelle circensi, settori che rischiavano di rimanere emarginati se si fosse proseguito con l'impianto originario della legge delega sul cinema.

Le audizioni hanno consentito anche di mettere a fuoco le criticità del settore ed è su queste che si è ritenuto opportuno lavorare. Sono emerse criticità diverse per i vari settori e generi dello spettacolo. Do atto anche alla relatrice dello spirito di apertura al confronto e di collaborazione nell'affrontare le proposte pervenute da tutte le componenti, anche di minoranza, che hanno portato al testo definitivo, che risponde, se non a tutte, sicuramente alla maggior parte delle problematiche emerse. Rispetto a quello originario, il testo licenziato dalla Commissione presenta significative integrazioni in risposta a un settore che attende una riforma organica da qualche decennio. È del 1985, infatti, la legge n. 163, istitutiva del FUS, che aveva lo scopo di ricondurre a un quadro unitario il sostegno statale ai diversi settori dello spettacolo, disciplinato da specifiche e numerose leggi. A questa legge di carattere generale non è seguita però la riforma organica dei diversi settori prevista dalle stesse disposizioni transitorie. Tale riforma, prevista da più di trent'anni, non ha fino a oggi ancora trovato attuazione. Vado a sottolineare alcuni aspetti importanti di questo disegno di legge. Si tratta di una legge delega, ma non di una delega in bianco al Governo. Il provvedimento in esame contiene una serie di principi e di criteri direttivi precisi e ben definiti, per cui i decreti legislativi che seguiranno dovranno mirare innanzitutto all'ottimizzazione e alla semplificazione, anche con l'abrogazione di precedenti disposizioni frammentarie e disorganiche, che negli anni di attesa del provvedimento quadro hanno lasciato molto spesso spazio alla gestione casuale e contingente delle iniziative. Anche gli interventi economici a sostegno della promozione e della realizzazione delle iniziative e degli enti attuatori, pur fondamentali, sono stati gestiti per lo più al di fuori di un quadro organico e strategico. Un secondo aspetto è nell'obiettivo del rilancio e dello sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue varietà, comprese quelle di più recente affermazione, che altrimenti rischiavano di rimanere escluse e di nuovo prive di adeguato riconoscimento e sostegno. Ne beneficiano la musica contemporanea popolare, la danza, i carnevali storici e le rievocazioni storiche che, oltre al riconoscimento giuridico, avranno per la prima volta la possibilità di accedere al FUS, in quanto parte integrante del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese. Una terza considerazione riguarda l'aumento progressivo delle risorse destinate alla dotazione del FUS, che sarà ripartito con nuovi criteri strategici e comprendenti anche i nuovi settori. Il FUS disporrà di una dotazione di ulteriori 9,5 milioni di euro per il 2018 e il 2019, che diventeranno 22,5 milioni a decorrere dal 2020. Per il riparto dovranno essere seguiti criteri di valorizzazione della qualità delle produzioni; di finanziamento selettivo per i progetti dei giovani *under* di conservazione del patrimonio musicale, teatrale e coreutico; di promozione dell'accesso al credito agevolato, con un particolare riferimento ai giovani artisti; di piani straordinari per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture destinate allo spettacolo, con particolare riferimento ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, ai Comuni di minori dimensioni, quelli su cui maggiormente ricade la limitatezza di risorse destinate alla cultura. Positivo è che il FUS venga destinato per almeno il 3 per cento alle scuole di ogni ordine e grado per la formazione, puntando a creare un sistema virtuoso che, tramite la formazione e l'educazione allo spettacolo dal vivo, porti sul lungo periodo un pubblico maggiore, più qualificato e sensibile; un investimento, dunque, per il futuro. L'articolo 2 al comma 3 si dedica alle criticità finanziarie in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche. Nel corso di questa XVII legislatura sono intervenute molte disposizioni volte a fronteggiare la crisi del settore lirico-sinfonico, prevedendo il riassetto della *governance* delle fondazioni e relativi piani di risanamento ed erogando risorse che ne hanno consentito la sopravvivenza. In particolare, cito la legge Bray, che ha previsto la possibilità di accedere a un fondo speciale di 75 milioni di euro e la concessione di finanziamenti fino ad un massimo di trent'anni. Si è trattato, però, di un provvedimento tampone che ha consentito la sopravvivenza per quelle fondazioni che, versando in condizioni di gravissima difficoltà economica, hanno ritenuto di farvi ricorso. Ora vengono previsti nuovi criteri per l'attribuzione del FUS e una nuova disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Nello specifico, si prevede lo scorporo dal FUS delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni e lo spostamento al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari. Altra sottolineatura voglio fare all'estensione dell'Art bonus all'intero settore dello spettacolo. Il credito d'imposta del 65 per cento per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, già oggi applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, è esteso anche alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo senza scopo di lucro. strumento, quello dell'Art bonus, che si sta rivelando veramente strategico per dare nuovo apporto di risorse finanziarie al mondo dello spettacolo e della cultura in generale; Art bonus nato per sostenere le erogazioni liberali destinate a interventi su beni monumentali di proprietà pubblica, ma che è bene venga esteso anche alla realizzazione di attività nel campo culturale. Per assicurare una corretta e sistematica valutazione sull'efficacia degli interventi e indirizzare le politiche del Ministero, viene istituito, analogamente a quanto previsto dalla legge sul cinema, ma con gli opportuni adattamenti dovuti alla specificità del settore, il nuovo organismo del consiglio superiore dello spettacolo.

dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, estendendo a tutte le attività di spettacolo la semplificazione amministrativa attualmente prevista solo per le attività circensi e di spettacolo viaggiante. È un tema delicato, sul quale sono intervenuto anche in fase emendativa. Molti degli spettacoli ingiustamente definiti minori - ingiustamente perché rappresentativi della cultura e delle tradizioni popolari, quelle diffuse sul territorio - vengono realizzati solo per la grande passione e grazie all'attività volontaria di molti appassionati: il popolo delle *pro loco* e delle associazioni di volontariato. Consentitemi di definirli popolo, proprio perché costituito da una moltitudine di persone che operano solo per la loro grande passione. Ricordo che il testo unico sullo spettacolo risale al 1931 - è un regio decreto ed è tuttora il riferimento normativo base a cui si ispirano i successivi provvedimenti che regolano l'organizzazione di eventi di varia natura. Certamente non dobbiamo non ricordare gli incidenti che si sono verificati, come quello di Torino del 3 giugno. Io vengo da una provincia dove il 2 agosto di tre anni fa, durante una festa popolare, a causa di una inondazione del tutto imprevedibile sono decedute quattro persone. Non dobbiamo sottovalutare nemmeno il rischio attentati, che, se non hanno per nostra fortuna colpito l'Italia, hanno interessato altri Paesi; rischio che ha ispirato recenti circolari del Ministero dell'interno, volte al potenziamento delle misure di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche.

vorrei svolgere una considerazione su un tema, forse l'unico, che ha sollevato, per diversi aspetti e a seconda delle sensibilità individuali, considerazioni e posizioni diverse, talvolta nettamente contrapposte: quello relativo all'utilizzo degli animali nei circhi. L'abbiamo constatato anche durante il dibattito d'Aula. Riteniamo che in questo caso la delega affidata al Governo, senza indicazione di tempistiche, consenta un'ulteriore approfondita analisi delle diverse tesi, cercando, laddove possibile, la mediazione tra le diverse sensibilità, quella di chi nei circhi lavora, anche con gli animali, e che legittimamente difende il proprio lavoro e quella di chi invece ritiene che questo tipo di lavoro debba essere esercitato senza l'impiego di animali. In questo interventi mi sono limitato a sottolineare solo alcune delle principali caratteristiche del disegno di legge che è sottoposto al voto dell'Assemblea; la vastità e la complessità dei temi affrontati, d'altronde, non consentivano di fare altrimenti. Un testo condiviso dal Gruppo di Alternativa Popolare, che lo voterà con convinzione.

ma sicuramente sarebbe stato utile evitare una nuova, ennesima delega al Governo e magari investire risorse vere. I tagli alla cultura in questi anni sono stati pesanti e non indolori hanno modificato non poco il variegato mondo culturale e dello spettacolo. Questi tagli non sono stati fatti solo dai Governi di destra, da quelli che "con la cultura non si mangia", ma sono proseguiti anche in questa legislatura.

Il nuovo regolamento per accedere ai fondi del FUS aveva creato aspettative, ma poi sono arrivate le conferme dai numeri. Infatti siamo dinanzi al sostanziale definanziamento del FUS nel triennio 2017-2019:

che prevedete con questa legge per il 2018-2019 e i 22 che prevedete per il 2020 non riescono a far raggiungere al FUS, al FUS, nella migliore delle previsioni, nemmeno l'ammontare del 2016. Quindi i numeri ci riportano alla cruda realtà. Questi dati sono così reali che non possono essere cambiati nemmeno dal trionfalistico *storytelling* di questa legge. Non basta fare un provvedimento organico, come ci è stato detto negli interventi di maggioranza, per allargare l'accesso al FUS a chi ne è stato fin'ora escluso, se poi non vengono aggiunte risorse. Il mondo dello spettacolo e della cultura si muove in un quadro molto difficile, al punto che l'accesso alla cultura del pubblico è un serio problema. Non è un caso che aumenta la partecipazione dei cittadini agli eventi gratuiti, quelli ovviamente promossi dal Ministero e da alcuni grandi Comuni. In un periodo di grave crisi occupazionale e riduzione del potere d'acquisto, i consumi culturali vengono tagliati, ma appena è possibile i cittadini cercano di soddisfare la loro curiosità curiosità culturale e intellettuale partecipando a ogni incontro gratuito. Sono in aumento le nuove forme di partecipazione e autorganizzazione dei cittadini e degli operatori culturali a sostegno delle forme d'arte del contemporaneo. Le occupazioni culturali di cinema e teatri, l'apertura di nuovi spazi associativi dedicati alla cultura, il fiorire di progetti di *coworking* spesso legati ad attività creative e culturali sono il segnale che questo mondo ha la forza per ripensarsi e trovare nuovi modelli di *governance* e sostenibilità perché troppo spesso esclusi da finanziamenti e sostegni pubblici. Anche il terzo settore culturale si rinnova e cerca una terza via tra associazionismo e impresa culturale, ma nemmeno questa volta abbiamo riconosciuto e previsto interventi innovativi fiscali e di maggiore efficienza per alcuni strumenti fondamentali per il funzionamento di questo mondo.

risorse. Non basta raccontare che si approvano leggi che da tempo si aspettano, se poi non si fanno scelte conseguenti e non si investono risorse. Si è cercato di mascherare i tagli alla cultura annunciando l'arrivo di finanziamenti da parte di privati che, a parte quelli per i grandi eventi, in realtà non sono arrivati. Ieri il Ministro ha parlato di 180 milioni provenienti dall'Art bonus*,* ma nello stesso tempo vi siete rifiutati di approvare un nostro emendamento in cui si specificava che le risorse private sono da considerare aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti pubblici. Si tratta, dunque, di un alibi per il definanziamento pubblico. di legge in esame separa le fondazioni liriche, rispondendo ad una richiesta che da sempre chi si occupa di spettacolo ha fatto alla politica. Si ritorna però al dunque: e le risorse aggiuntive? Siamo al quarto intervento legislativo in questi in questi anni su fondazioni liriche e sono ancora molti i nodi aperti. In questi anni le pessime scelte della politica e dei sovrintendenti sono state pagate con il taglio di posti di lavoro e bilanci insostenibili. È bene che ci siamo posti l'obiettivo di riconoscere le responsabilità, ma sappiamo bene che nella frase: «le responsabilità accertate» può nascondersi un inganno senza fine. In questi anni la politica ha preferito fare altre scelte anche dinanzi all'evidenza.

avremmo dovuto affrontare alcuni nodi, come ad esempio (ne abbiamo parlato spessissimo in Commissione durante le audizioni) quello della ricostituzione dei corpi di ballo dipendenti dalle fondazioni liriche e di tutte le attività tipiche che in questi anni sono state esternalizzate, facendo rientrare al lavoro i lavoratori che attualmente sono dipendenti di ditte in appalto. Il pareggio di bilancio è uno degli obiettivi, ma non può mortificare l'attività delle fondazioni liriche e le capacità artistiche e tecniche di cui il nostro Paese è particolarmente ricco, perché è positivo far quadrare i conti, ma è anche bene dire una volta per tutte che bisogna investire in cultura. Da anni poniamo il problema della stabilità dei posti di lavoro proprio per valorizzare quelle competenze tecniche, artigianali e artistiche che rappresentano esperienze uniche per il nostro Paese e che devono essere salvaguardate mantenendole - ripeto - all'interno dei teatri, creando un sistema proprio per valorizzare il lavoro. Le risorse devono essere pubbliche e non solo dello Stato: servono risorse vere delle Regioni e degli enti locali.

la graduale dismissione avrebbe consentito consentito anche un reale rinnovamento della proposta delle attività circensi perché i dati ci dicono che negli ultimi anni anche il circo è sottoposto ad una crisi complessiva di partecipanti agli spettacoli. Quindi sarebbe stata anche l'occasione per

per metterci in sintonia con le sensibilità dell'opinione pubblica, proprio come ha detto ieri il Ministro nella sua replica. Invece è mancato il coraggio. Avete preferito una lettura del Paese che volge lo sguardo indietro, avete preferito formule vaghe per prendere impegni generici. Il dibattito ascoltato spesso è stato surreale, pregiudiziale e di posizionamento, rivelando in molti interventi, devo dire, anche poca conoscenza del merito. Non si sono scontrati due estremismi ma due visioni diverse,

di questo provvedimento perché i vaghi impegni presi per i decreti attuativi saranno per noi motivo per proseguire questo lavoro e questa battaglia, perché vogliamo guardare al futuro anche delle arti dello spettacolo, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo di tradizioni e delle arti circensi.

non ci è capitato spesso di sperimentare nel corso di questa legislatura dai banchi dell'opposizione. Poi vorrei fare qualche considerazione generale anch'io sul testo, specificando che anche anche noi avremmo preferito che non avesse la forma di una delega, anche se il caso del riordino di una materia così ampia forse trova un qualche un qualche barlume di giustificazione in più rispetto alla marea di deleghe con le quali siamo stati inondati nel corso di questa legislatura. Ci auguriamo, però, che i decreti attuativi che seguiranno alla delega non facciano la fine né dei decreti attuativi conseguenti alla cosiddetta buona scuola né di quelli conseguenti alla legge di riordino del settore cinema che ancora ci pare navighino nel porto delle nebbie. Devo dire che il Movimento 5 Stelle, come forza di opposizione, molto ha contribuito, durante i lavori di Commissione e di Aula, all'esame di questo testo e anche al "restringimento", all'apposizione di paletti ad una delega che era veramente tanto, tanto ampia all'origine. Vorrei fare anche una considerazione sullo spettacolo dal vivo in generale, perché va benissimo questo tentativo di riordino della normativa in materia per renderla più organica e più efficace e va benissimo trovare nuove forme di sostegno come l'Art bonus esteso allo spettacolo dal vivo anche se, come ha rilevato prima di me la collega Petraglia, non vorremmo che questa misura mascherasse poi la volontà di demandare al privato il sostegno di questo settore si riducessero sempre di più gli interventi pubblici a sostegno. Vanno bene anche le risorse fresche che sono state trovate, anche se poi in realtà il Fondo ha un'entità tale da poter costituire un vero sostegno. Però ricordiamoci che bisogna mantenere anche gli impegni per inserire nelle scuole attività tese alla promozione delle arti e allo sviluppo di una sensibilità e di una passione che sono fondamentali per creare una società non solo intellettualmente e culturalmente più elevata, ma anche fruitrice e, così facendo, creare nuovo pubblico. Parallelamente si poteva cogliere l'occasione, con un nostro emendamento, per approvare la nostra proposta di riduzione dell'IVA sulla bigliettazione. Sappiamo, infatti, che questo sarebbe andato sicuramente a beneficio di una maggiore frequentazione dei luoghi della cultura non solo da parte dei giovani e degli studenti, ma anche da parte degli adulti,

proposta di istituire un tavolo programmatico per promuovere l'inserimento dello spettacolo dal vivo nei programmi turistici, pratica che, in realtà, c'è già, ma non è coordinata e non è efficace, ossia tale da garantire un circuito turistico che prenda in considerazione anche lo spettacolo dal vivo come forma di attrattiva per i turisti che vengono a visitare il nostro Paese

della senatrice Blundo; anche se, rispetto alla danza, permane la nota fortemente critica che, a fronte della delega alla ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo e alla promozione della produzione artistica e della sperimentazione, abbiamo paradossalmente, nella realtà, lo smantellamento di un corpo di ballo, quello dell'Arena di Verona, la chiusura di compagnie storiche e il fatto che progressivamente si è arrivati in Italia ad avere solo due corpi di ballo stabili: quello della Scala di Milano e quello del Teatro dell'Opera di Roma. Ci chiediamo dove andranno poi tutti questi nostri giovani che vorranno intraprendere la carriera di danzatori se in Italia non abbiamo un bacino di assorbimento di tutti questi talenti. Del resto anche il nostro Bolle dice che la danza rimane ignorata e maltrattata in Italia. Nel campo delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Movimento 5 Stelle molto si è battuto per rivedere il sistema di controllo sulla gestione economico-finanziaria e artistica delle fondazioni, perché la *mala gestio*, finora, ha avuto ripercussioni solo sulle masse artistiche e tecniche. Siamo riusciti a far introdurre tra i criteri per l'assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo la responsabilizzazione del sovrintendente per la gestione economica e finanziaria e anche la considerazione dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente, con la speranza che questo porti ad avere una maggiore qualità, ma soprattutto che porti all'eliminazione del famigerato algoritmo. Infine, siamo riusciti a ottenere in Assemblea il cosiddetto Daspo per i sovrintendenti che dimostreranno di non aver saputo gestire bene e accuratamente da un punto di vista economico e finanziario le fondazioni e che quindi non potranno più essere rinominati per ricoprire lo stesso ruolo all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Siamo anche riusciti a inserire un pezzettino di una risoluzione che abbiamo fatto approvare all'unanimità un paio di anni fa: la cosiddetta mappa dell'abbandono. Nel testo infatti

l'iscrizione o l'abbonamento a scuole di danza, di musica o di teatro per i giovani tra i cinque e i diciotto anni e spero davvero che in legge di stabilità questo impegno sia onorato; noi tutti ci impegniamo affinché il Governo trovi queste risorse. Passiamo alle note dolenti. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche siamo rimasti fermi al palo della selezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici con bandi pubblici anche internazionali; e dire che il Ministro è così affezionato a questi bandi pubblici anche internazionali, ma evidentemente, in questo settore, sono altre sono altre le logiche che prevalgono. È rimasto al palo anche il conflitto d'interesse per i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, oltre che per i sovrintendenti e i direttori artistici. Quindi, anche qui continueranno a perpetrarsi quelle quelle dinamiche per cui talvolta, a seguito di questi conflitti d'interesse, forse non canterà il miglior tenore o la migliore soprano in uno spettacolo o forse saranno acquistati degli allestimenti che probabilmente potevano non essere acquistati, nonché materiali e quant'altro. Per quanto riguarda i teatri nazionali, ci dispiace molto che non siano passate le nostre proposte di riordino della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento delle scuole di teatro, dato che sono tante, molte non regolamentate, a scapito della qualità della formazione, quindi anche del nostro buon nome in quei settori a livello nazionale e internazionale. Ci dispiace che non sia stata presa in considerazione neanche la proposta di revisione di modalità di nomina degli incarichi dirigenziali, per le stesse motivazioni per cui tanto c'eravamo battuti per le fondazioni lirico-sinfoniche. Anche il consiglio superiore per lo spettacolo, a nostro avviso, è un organismo destinato a lavorare nell'opacità, perché la nostra proposta di trasparenza sulle nomine e sui lavori non è stata accolta, come non è stata accolta la selezione, anziché la nomina, dei suoi componenti. Infine, non c'è nulla di concreto per il riconoscimento giuridico professionale dei lavoratori del settore né per il trattamento previdenziale. Invece, si è data giustificazione normativa alla mobilità. Concludo con tre punti ancora critici. Non è stato fatto nulla e non sono state accolte le nostre proposte per porre rimedio al fenomeno del *secondary ticketing*. È stato fatto un timido tentativo, con l'approvazione di un emendamento, sul progressivo abbandono della bollinatura SIAE sui dispositivi musicali, ma nulla si è fatto per sanare la situazione in cui ancora oggi la SIAE opera, di effettivo monopolio, a dispetto di una direttiva comunitaria che invece ci impone di fare altro. Infine, non è stato ascoltato il mondo dello spettacolo viaggiante e abbiamo assistito a una clamorosa retromarcia sull'utilizzo degli animali all'interno delle attività circensi. Per tutte queste ragioni, valutando il fatto che ci troviamo al primo passaggio parlamentare e che questo provvedimento approderà alla Camera, noi esprimeremo un voto di astensione, unicamente perché speriamo che durante l'esame da parte della Camera ci sia ancora la buona volontà per fare uscire da questo Parlamento il miglior testo possibile.

Ringrazio anch'io la relatrice Di Giorgi per l'impegno che ha profuso per migliorare un testo che era arrivato in Commissione molto diverso. Sono il primo a riconoscere i miglioramenti apportati a un articolato prima pletorico, ripetitivo e poco concreto. Tuttavia, abbiamo scelto, come Forza Italia, di sospendere il nostro giudizio perché purtroppo questa legislatura, come ho già ricordato in discussione generale, verrà ricordata come la legislatura dei voti di fiducia e delle deleghe assegnate Il dibattito sul codice per lo spettacolo è stata anche l'occasione per promuovere una ricostruzione storica dell'intervento pubblico amministrativo, di Governo e parlamentare in favore della cultura. Il Ministro, ieri in Aula, ha avuto la cortesia di ammettere che i risultati conseguiti da questo Governo sono il frutto di un lavoro nato da lontano.

Letta, poi Renzi, oggi Gentiloni Silveri. Siamo molto diversi perché noi per lo spettacolo dal vivo non abbiamo esercitato una delega nel 2010, ma abbiamo proposto alle Commissioni di merito, prima, e all'Assemblea, dopo, una legge di sistema dove c'era scritto tutto. Non abbiamo delegato il Governo a fare, dopo, la sua cucina nelle segrete stanze del palazzo. Abbiamo affrontato le Commissioni di Camera e Senato e l'Assemblea con una seduta notturna, chiedendo il voto. Potevamo anche pretendere il voto di fiducia, che è l'*extrema ratio* per approvare un provvedimento controverso. No, noi abbiamo invece affrontato, se non ricordo male, circa venti ore di seduta continua,

all'articolo 2, comma 1, non si parla di codice dello spettacolo, ma delle fondazioni lirico-sinfoniche. Lo stesso Governo nel testo che ci ha proposto e che la Commissione ha approvato ammette subito, all'articolo 2, comma 1, che il vero problema sono di nuovo le fondazioni lirico-sinfoniche, nuova delega al Governo per scrivere altri decreti legislativi attuativi in merito alla legge n. 160 del 2016, sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Nel secondo periodo - sempre del comma 1 e sempre dell'articolo 2 - si fa riferimento alla delega per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti,

Prima il bubbone, le fondazioni lirico-sinfoniche: delega per attuare la famosa legge n. 160, quindi niente di nuovo sotto il sole.

citati. I criteri adottati sono generici: favorire la promozione internazionale delle opere e dello spettacolo italiano, aiutare i giovani, favorire la cittadinanza, l'integrazione culturale, il credito agevolato, l'accesso della disabilità nello spettacolo, l'associazionismo, la musica popolare contemporanea la partecipazione del privato, il 3 per cento per le scuole di ogni ordine e grado. Tutti principi importanti, che sono però tutta poesia. La verità è data dalla distribuzione dei fondi esistenti, che vengono implementati fino a 22,5 milioni di euro nell'anno del signore 2020. Quindi noi abbiamo un grande stanziamento che raggiungerà la capienza di 350-360 milioni e bisogna decidere come spendere tutti questi soldi.

prerogativa delle autorità di Governo decidere e pianificare, devono essere concertati con le Regioni in sede di conferenza unificata. C'è quindi una più stringente collaborazione con le Regioni. Si tratta di un elemento importante.

la prevalenza sia nelle strategie del Governo, sia nella spesa che il Governo, l'amministrazione centrale e le Regioni dovranno sostenere per favorire lo spettacolo in Italia.

e l'autonomia di tutte le fondazioni ed avevamo imposto alle stesse di aderire al contratto nazionale di lavoro e di eliminare tutti quei contratti integrativi aziendali che avevano prodotto una miriade di privilegi che erano assolutamente ingestibili e che avevano lasciato sul terreno oltre 300 milioni di debiti. Oggi mi accorgo che questi debiti faticano ad essere riassorbiti, che il Governo ci chiede un'ulteriore delega e che addirittura nell'ordine del giorno del

Cito Bondi: «Se non fossimo intervenuti, davvero avremmo lasciato perire l'opera lirica in questo Paese. Ho proposto questo provvedimento per salvare l'opera lirica, non per metterla in difficoltà. Non ho mai considerato questo provvedimento come chiuso al confronto e blindato, anzi» - e l'ho ricordato, siamo andati in Aula - «l'ho sempre considerato un provvedimento legislativo aperto» (non una delega) «non solo al confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione, ma anche, fuori da quest'Aula, con le organizzazioni sindacali». Quindi noi siamo molto diversi da questo Governo. Concludo dicendo al ministro Franceschini che non mi voglio paragonare a lui, perché non posso dimenticare - e voglio richiamare l'attenzione dei miei colleghi che Franceschini, oggi Ministro della cultura, che sta facendo la riforma del Ministero attraverso atti amministrativi, depotenziando le sovrintendenze, che ha fatto la riforma del cinema con una delega e sta facendo la riforma della spettacolo con una delega, è lo stesso uomo che, Capogruppo del PD, PD, chiese nell'Aula della Camera dei deputati le dimissioni del ministro Bondi dopo i fatti di Pompei. Pompei oggi rinasce perché il Governo Berlusconi ed il ministro Bondi hanno sviluppato una grossa attività di recupero ottenendo 110 milioni dall'Unione europea, grazie ai quali i Governi successivi hanno aperto 35 cantieri che hanno salvato Pompei. *(Applausi del senatore Floris).* Quindi, noi non facciamo demagogia sulla cultura, non chiediamo le dimissioni del ministro Franceschini per i crolli a Pompei, che sono continuati. Siamo persone serie, ci confrontiamo nelle Commissioni; non chiediamo deleghe, andiamo in Aula, ci mettiamo la faccia *(Applausi del senatore Floris)* e approviamo i provvedimenti che riteniamo opportuni per salvare davvero - e non per finta - tutto e non parte dello spettacolo in Italia. Per tutte queste motivazioni, esprimeremo su questo provvedimento un voto di astensione. *(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quest'Assemblea sta per votare un disegno di legge che si occupa di cultura in una legislatura che, per fortuna, è stata molto ricca di provvedimenti e - aggiungo - di finanziamenti per un settore vitale del nostro Paese. Dico «per fortuna», ma in realtà si tratta di una precisa volontà politica. In questo caso esaminiamo il disegno di legge delega sul codice dello spettacolo, che, come ricorderete, fu stralciato dalla legge sul cinema e oggi trova finalmente attuazione dopo circa trent'anni di attesa. Uno stralcio, benché criticato da molti colleghi, opportuno e utile, voluto dal Senato della Repubblica perché c'era bisogno di andare nel dettaglio delle deleghe che conferivamo al Governo, e la dialettica all'interno della Commissione e del Parlamento in generale credo abbia dato buona prova di sé. Un provvedimento particolarmente virtuoso, secondo noi, perché il Parlamento ha esercitato, questa volta davvero fino in fondo, il suo ruolo. Nella 7a Commissione, che mi onoro di presiedere, sono stati sono stati auditi una quarantina tra personalità e associazioni del settore, per recepire le volontà degli operatori, capirli, comprenderne le necessità. Sono stati poi discussi, e in molti casi approvati, emendamenti e pareri di senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. Un lavoro importante che ha dato i suoi frutti, in questo disegno di legge composto da sette articoli, che nasce con l'obiettivo di dare supporto allo spettacolo dal vivo, che noi riteniamo essere una grande ricchezza per il nostro Paese. Voglio sottolineare uno dei passaggi che mi appare più significativo: quello che riguarda la definizione del Fondo unico per lo spettacolo. il FUS era unico; con questo provvedimento si distingue tra le risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e le risorse destinate a tutto il resto del mondo dello spettacolo. Questo serve a fare chiarezza e a dare equilibrio e responsabilità agli operatori, incluse, e forse soprattutto, le fondazioni lirico-sinfoniche. Viene poi riconosciuto il valore educativo e formativo dello spettacolo, con interventi specifici per la scuola: il 3 per cento del FUS andrà alla scuola con un accordo preciso, perché gli spettatori di domani vengono formati sui banchi di scuola. Insieme a 18App, questo testimonia di quanto si crede nei giovani codice dello spettacolo per la prima volta riguarda anche i carnevali e le rievocazioni storiche, ammessi all'erogazione del FUS. È il coronamento di una battaglia, anche personale, per riconoscere dignità culturale e valore economico a manifestazioni tipiche tipiche del nostro Paese e che contribuiscono alla specificità italiana e alla produttività di tante economie locali. All'inizio dicevo che questo è solo l'ultimo di tanti provvedimenti che i Governi, Renzi prima e Gentiloni Silveri oggi, hanno definito e finanziato. Voglio solo ricordare i più importanti: la legge sul cinema con la creazione di un fondo di 400 milioni, con il potenziamento delle sei misure che riguardano il *tax credit*; l'introduzione nella legge di bilancio del 2015 nella legge di bilancio del 2015 del *bonus* da 500 euro per i consumi culturali dei neo maggiorenni. Una misura importante - tra l'altro avviata nuovamente per la seconda annualità proprio in questi giorni - che riguarderà anche tutti coloro che compiranno diciotto anni il prossimo anno. È stata usata da una platea dell'80 per cento degli aventi diritto e ha riguardato prevalentemente l'acquisto di libri. Un passaggio importante, e rispetto ai decreti attuativi ministeriali della legge sul cinema

Nuovi fondi per la tutela del patrimonio e i grandi progetti culturali: 150 milioni di euro nel 2016, 170 milioni nel 2017; fondi in crescita. La senatrice Petraglia ha detto che in questi anni i fondi per la cultura in Italia sono stati drammaticamente tagliati, ahimè non è vero: con questi Governi e grazie a questo Parlamento, negli ultimi anni i fondi per la cultura sono aumentati e anche in maniera consistente,

Vogliamo ricordare poi l'Art bonus, che ha reso permanente il credito d'imposta del 65 per cento per il finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali, per il sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, per le fondazioni lirico-sinfoniche, per i teatri di tradizione, nonché per la realizzazione, il restauro e il potenziamento di strutture e di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo, esteso proprio con il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi a tutte le forme di spettacolo e quindi anche ai festival

dello spettacolo e di supportarle nelle forme e con la libertà necessarie, e lo facciamo dando loro un'importante agevolazione fiscale. È un invito a tutto il Paese a credere nelle nostre attività culturali. Concludo questa sintetica carrellata con il provvedimento che ha reso autonomi 20 grandi musei italiani, con il bando internazionale che ha selezionato 13 italiani, tre tedeschi, due austriaci, un britannico e un francese alla loro direzione e che sta dando ottimi risultati: lo posso dire anche a seguito della recente visita, svolta

come delle opposizioni. Oggi, ad esempio, a proposito della questione relativa alla SIAE, è stato introdotto un piccolo passaggio importante che faciliterà gli operatori culturali su tutto il territorio.

una risposta seria alle giuste aspettative dei lavoratori della cultura, che da troppo tempo aspettano la corretta tutela dei loro diritti: delega va esattamente in questa direzione e siamo molti orgogliosi di averla scritta. È un atto politico chiaro, che segue una giusta traccia di continuità, che fa della cultura una priorità assoluta dell'attività di Governo. è cultura, è attività culturale e produzione culturale: avevamo il dovere di occuparcene nella nostra veste istituzionale e sono quindi orgoglioso del lavoro svolto insieme e sono felice di annunciare il convinto voto favorevole al provvedimento in esame.

titolo: «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia». *(Segue la votazione).*

enti locali. Il disegno di legge può sembrare irrilevante, ma è estremamente significativo. Noi trattiamo della volontà di una comunità municipale di passare dalla dalla Regione di appartenenza a un'altra Regione,

hanno la possibilità di determinare trasferimenti erariali in maniera diversa dalle Regioni a statuto ordinario: hanno, insomma, una possibilità diversa di interlocuzione con gli enti locali. Noi, ancora una volta, pur avendo adesso una piccola "patata calda" tra le mani, non vogliamo affrontare il grande tema del governo del territorio, della frantumazione del governo del territorio in un numero a mio giudizio eccessivo di Comuni e di Regioni, e il grande tema della continuità dell'esistenza di Regioni a statuto speciale. Per Per questo motivo ho chiesto d'intervenire: non tanto per avanzare giudizi sulla comunità di Sappada, che legittimamente utilizza le previsioni normative per potere meglio decidere della sua collocazione istituzionale, ma perché quest'Assemblea e il Parlamento in generale continuano a rifiutarsi di affrontare il grande tema del governo del territorio e, soprattutto, degli enti locali. tema che avevo chiesto venisse affrontato quando abbiamo discusso della riforma costituzionale; richiesta che è stata respinta dal Governo e dalla maggioranza come parte non essenziale di una riforma costituzionale. Ritengo, invece, che la riforma del governo del territorio sia l'argomento principe di una possibile riforma costituzionale, perché il nostro Paese, che viene additato come uno dei Paesi che impiega maggiori risorse nel mantenere un apparato politico e burocratico parcellizzato sul territorio, non può, a mio giudizio, continuare nel tempo a sostenere i costi di una così elevata parcellizzazione e di una così difforme autonomia degli enti locali e delle Regioni nell'ambito dello stesso contesto nazionale. La nostra, purtroppo, ormai non è più una Nazione ma è un agglomerato di Regioni: di fatto ventuno (troppe), assolutamente in numero esorbitante, tutte tra loro scollegate e tutte tra loro in grado di trattare in maniera diversa i rapporti con i Comuni e con gli enti locali, tant'è che nascono questo tipo di richieste. ripeto- assolutamente legittime dal punto di vista dell'impianto normativo del Paese, ma sulle quali noi ci dobbiamo interrogare. Non possiamo non interrogarci del perché un Comune chieda di passare da una Regione all'altra e, in questo particolare caso, da una Regione a statuto ordinario a una Regione a statuto speciale. Non possiamo non interrogarci del perché nel nostro Paese le fusioni volontarie volontarie tra Comuni siano ancora così poche; del perché gli strumenti di incentivazione della semplificazione amministrativa in tema di Governo locale non esistano;

di fortuna per il cittadino il nascere in un Comune o in una Regione piuttosto che in un'altra per la diversità del trattamento che può ricevere a seconda del suo luogo di residenza o di nascita.

passerà. Ripeto, esso rientra nell'assoluta legittimità dell'impianto normativo del nostro Paese e, quindi, è una richiesta che abbiamo il dovere di esaminare. Naturalmente non ci interroghiamo sul perché in queste ore una situazione molto più complessa e sicuramente più profonda, come l'indipendenza della Catalogna, sia oggetto addirittura di arresti da parte del Governo spagnolo, solo per evitare il *referendum* sulla separazione Non ci interroghiamo, ma continuiamo a tenere in piedi un Paese ormai disgregato dal punto di vista istituzionale. La nascita delle Regioni a statuto speciale aveva una sua logica nell'immediato Dopoguerra ed ha avuto anche una sua logica in alcuni episodi legati all'esistenza

essere composta da realtà sempre più ampie e sempre più omogenee, è difficile continuare a pensare a questi impianti. A meno che non si voglia pensare che l'Europa delle cosiddette regioni sia poi finalizzata, nel senso che abbia come sbocco finale la possibilità di non essere più l'Europa delle Nazioni, ma di essere solamente l'Europa dei territori. Spero che queste mie

solamente l'aspetto organizzativo, ma anche i principi fondamentali della Repubblica. Bisognerebbe chiarire esattamente cosa noi intendiamo per federalismo, ove mai se ne continui a parlare, visto che mi pare una parola un po' andata in decadenza,

una riforma delle Province che grida vendetta al cospetto di Dio, oltre che degli uomini. Pur avendo approvato l'ordine del giorno Ranucci, durante il dibattito costituzionale, non volete entrare nell'ottica della revisione dell'impianto delle Regioni, perché è quello il punto dolente, anche dal punto di vista del bilancio del Paese. Noi abbiamo ventuno entità fuori controllo: fuori controllo nella spesa, fuori controllo nella dinamica e nella qualità di questa spesa. Continuiamo, nello stesso Mezzogiorno d'Italia, ad avere la parcellizzazione dei fondi europei per Regioni; quindi non si fanno grandi piani infrastrutturali che siano veramente interregionali. Queste cose non le dico solo io; prima di me le hanno dette anche illustri economisti dell'area della sinistra, come Nicola Rossi, che ha più volte lanciato l'allarme sul cattivo utilizzo dei fondi europei, in assenza di una strategia complessiva di territorio vasto. Da questi piccoli episodi, prendiamo spunto per un grande dibattito in ordine al riordino vero del governo del territorio del Paese, nell'ottica di ridurre i costi, migliorare i servizi e assicurare ai cittadini un trattamento egualitario, ovunque risiedano in questa nostra Nazione, perché siamo veramente in presenza di una diversità e di una disparità di trattamento nei servizi essenziali al cittadino, che credo non abbia pari in altre Nazioni d'Europa.

gran parte della popolazione friulana guardano ormai da molto tempo all'*iter* legislativo relativo al passaggio del Comune dolomitico alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Come ricordato dalla relatrice, l'*iter* istituzionale per il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia è stato avviato nel luglio del 2007, quando il Consiglio comunale della località montana deliberò l'indizione di un *referendum* consultivo. Tale *referendum* si svolse nei giorni 9 e 10 marzo 2008 e, a fronte della partecipazione di 903 elettori su 1.199 aventi diritto, il risultato fu di ben 860 elettori favorevoli, cioè il 95,2 per cento dei votanti, contro appena 41 voti contrari. Ricordo ancora che il 18 marzo 2009 il Consiglio provinciale di Udine approvò un ordine del giorno favorevole alla richiesta della cittadinanza di Sappada il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 23 novembre 2010, e quello del Veneto, il 28 giugno 2012, espressero medesimo parere favorevole. Questi, in estrema sintesi, sono stati i passaggi istituzionali di un *iter* ormai decennale, che nasce dal sentimento largamente diffuso nella comunità del Comune di Sappada di far parte dell'ambito amministrativo del Friuli, territorio verso il quale si sentono maggiormente affini e legati da profonde ragioni storiche e culturali. Sono passaggi e procedure che, a ben vedere, senza dubbio segnano l'espressione di una precisa volontà e il conseguente perseguimento di un ben definito obiettivo politico condiviso, che a mio avviso, signor Presidente, quest'Assemblea non può assolutamente negare. Ricordo ancora che Sappada è collocata nell'area geografica delle Dolomiti orientali, in quel territorio montano che si estende dalla Provincia di Belluno al Friuli, ed è proprio nel territorio montano del Friuli che si protende verso la Carnia che Sappada ha sempre trovato il suo naturale e storico punto di riferimento. Se dal punto di vista geografico e naturalistico sono evidenti i contatti con l'area friulana, anche sul piano storico i legami con il Friuli sono forti e radicati. il territorio di Sappada è stato legato a quello friulano sul piano amministrativo a partire dall'XI secolo, quando ai primi abitanti di Sappada, provenienti dal Tirolo, su invito dei conti di Gorizia, il patriarca di Aquileia concesse di poter risiedere in quel territorio dove ancora oggi vivono. Tale legame politico e amministrativo rimase intatto con la Repubblica di Venezia, a partire dal 1500, e, dopo una breve dominazione francese, si mantenne sotto il governo degli Asburgo. Solo alla fine dell'Ottocento la cittadina fu staccata dalla Provincia di Udine per passare a quella di Belluno. Tale passaggio, tuttavia, lasciò intatti diversi legami con il Friuli, a partire dall'appartenenza della parrocchia cittadina all'arcidiocesi di Udine. Merita infine ricordare come durante la Seconda guerra mondiale Sappada fece parte della Repubblica libera della Carnia, condividendo, anche in occasione della Resistenza e della lotta di Liberazione, il destino della vicina Carnia e del Friuli. tratto peculiare della comunità di Sappada è la lingua: i sappadini, infatti, parlano un dialetto germanico, il quale rappresenta il maggiore elemento identitario di quella comunità. Si tratta dello stesso tipo di dialetto di ceppo germanico parlato nelle comunità di Sauris e Timau nel Friuli-Venezia Giulia. Anche su questo piano, dunque, il passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia si configurerebbe come la naturale ricomposizione di una storica oasi linguistica che troverebbe ulteriori possibilità di promozione e tutela nell'ambito delle norme esistenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. È evidente, signor Presidente, come la richiesta dei cittadini di Sappada di ritornare nel loro naturale territorio del Friuli-Venezia Giulia sia il sentimento di una comunità che intende collocarsi nell'ambito territoriale e amministrativo che sente più proprio per ragioni storiche e culturali. Si tratta, dunque, di dare una risposta adeguata ad una richiesta del tutto fondata sul piano storico e culturale, come dicevo, che ha percorso tutto l'*iter* previsto dal dettato legislativo vigente in materia. Una richiesta, è bene ribadirlo, che ha ricevuto l'assenso, lo dicevo poco fa, dei Consigli regionali di entrambe le Regioni interessate: il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. che dare una risposta positiva in questo senso sia doveroso, tanto per la comunità di Sappada, che ormai da un decennio aspetta il raggiungimento di questo obiettivo, che per la montagna del Friuli che vedrebbe così ricomporsi quella naturale unità storica, culturale e linguistica che potrà essere uno dei fattori di possibile rilancio dello stesso territorio montano friulano, territorio del quale i cittadini di Sappada intendono far parte a pieno titolo. *(Applausi Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è costituito da un unico articolo che disciplina la procedura per il distacco del Comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli. Ovviamente la previsione contenuta nel testo in esame segue un *referendum* presso la locale comunità di Sappada che, in modo plebiscitario, ha scelto di aderire alla Regione con cui confina, lasciando la Regione Veneto, cui sinora appartiene, nel puntuale rispetto della previsione costituzionale in materia e delle procedure ad essa legate. Sappada è un piccolo comune - solo 1.317 abitanti - a ridosso della omonima cima, sulle prealpi Carniche, attraversato dal fiume Piave. Pochi giorni fa è assurta all'onore delle cronache perché sulla strada principale è passato il Giro d'Italia. La storia di Sappada, che parte nel X secolo, è tutta legata alla provincia di Udine, che lasciò nel 1853, per passare a quella di Belluno che poi, nel 1866, venne annessa all'Italia. Nel paese, che è una località a forte vocazione turistica cui sono legati molti miei ricordi d'infanzia, essendo a ridosso di un patrimonio ambientale straordinario, sono presenti anche tre differenti musei (Museo etnografico Giuseppe Fontana, Casa Museo della civiltà contadina e Piccolo Museo della grande guerra) e una grandissima varietà di iniziative culturali, artistiche e turistiche. Insomma, una realtà viva che, considerata la propria origine e la propria storia, si riconosce certamente di più nella realtà friulana che in quella veneta. Nella ricerca della propria tradizione e della propria cultura e nel riconoscimento di Sappada come isola linguistica germanofona è stato elaborato persino un vocabolario del dialetto sappadino, nato dall'esigenza di uniformare la scrittura del dialetto e di creare uno strumento alla portata di chiunque voglia consultarlo. Tantissime altre sono le iniziative culturali che evidenziano la ricerca delle proprie origini e la valorizzazione del proprio territorio. Tante sono le consuetudini e i modi di vita che i sappadini condividono con i friulani, oltre a condividerne il modello economico, il fiume e le montagne. La loro scelta va rispettata e, per noi che siamo parlamentari, onorata, considerato che la procedura prevede che debba essere il Parlamento a sancirla in modo ufficiale,

Dobbiamo, però, chiederci profondamente il perché di questa volontà, di questo desiderio di piccoli Comuni limitrofi a Regioni a statuto speciale quali il Friuli o la Provincia di Trento e Bolzano di richiedere quello che Sappada probabilmente otterrà. Certo: sanno che potrebbero offrire servizi migliori e in quantità superiori rispetto agli altri Comuni italiani che, in questi ultimi anni di Governi non eletti, si sono visti tagliare risorse e, nello stesso tempo, responsabilizzare ad erogare servizi e maggiori prestazioni per provvedimenti legislativi. Mi riferisco, ad

sempre con i fondi tagliati dal Governo centrale, dell'accoglienza dei migranti. Comunque, è giusto assecondare la volontà dei cittadini di Sappada, anche se, purtroppo, penso che ciò scatenerà l'invidia di molti Comuni vicini. *(Applausi

Signor Presidente, cari colleghi, prendo la parola su questo provvedimento rivolgendomi in primo luogo al Governo, al quale, in realtà, mi sono già rivolto nelle settimane scorse; e mi rivolgo al Governo ancorché si tratti di un provvedimento di iniziativa parlamentare (la cosa non mi sfugge). Mi sono rivolto al Governo con una corrispondenza indirizzata al Presidente del Consiglio, con la quale sollecitavo l'Esecutivo ad adoperarsi affinché questo provvedimento potesse essere ritirato. Se i passi che ho compiuto sono questi, va da sé che vi sono, da parte mia, sul disegno di legge in parola, delle riserve che ora cercherò di illustrare. Sono riserve che attengono a un profilo di carattere costituzionale e che sollevano e rimandano a questioni politiche, anche di carattere internazionale, su cui è bene che il Senato sia avvertito. Vengo alla questione di carattere costituzionale, precisando, in primo luogo, che non mi sfugge

che non vi è alcuna violazione del dettato costituzionale, né dello statuto della Regione Valle d'Aosta, nel provvedere a questo passaggio per il tramite di una legge ordinaria. Su quella sentenza vi fu una discussione dottrinaria di un certo interesse e intensità che io credo sia bene non trascurare. In ogni caso, ritengo che il Senato e poi la Camera, nel caso il provvedimento dovesse avere il disco verde da quest'Aula, e il Parlamento in generale è bene che si rendano conto della grande delicatezza istituzionale e costituzionale - e conseguentemente anche politica - della manomissione della manomissione della circoscrizione territoriale di una Regione a statuto speciale per il mezzo di un provvedimento legislativo ordinario. La prima grande critica che rivolgo a questo disegno di legge è il fatto che il passaggio viene provveduto attraverso una procedura legislativa ordinaria, anziché quella di carattere costituzionale con quattro letture.

che, quando è stato il Consiglio dei ministri ad assumere l'iniziativa legislativa per mandare avanti il passaggio di un Comune di una Regione ordinaria in direzione di una Regione a lo stesso Consiglio dei ministri si è cautelato - e non a caso - proponendo un disegno di legge di carattere costituzionale e non uno di carattere ordinario. Questo è accaduto in numerosi casi nel corso degli anni: degli anni: per Livinallongo, per Lamon e potrei citare altri casi ancora. Dobbiamo considerare che la casistica alla quale fare riferimento in queste vicende non è di uno o due Comuni; diciamo che c'è una lista d'attesa molto consistente, in particolare nella Regione Veneto, per il transito al Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento o di Bolzano. Dunque, tornando alla questione di carattere costituzionale, prudenza e attenzione

noi dobbiamo sapere che con un provvedimento di natura ordinaria si apre una porta di carattere procedurale che, nelle relazioni tra le Regioni ordinarie, le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e lo Stato, apre un percorso che si inizia ma oggettivamente non si sa dove e come può terminare. C'è una seconda questione. La motivazione per la quale la comunità sappadina decide di volersi ricongiungere al Friuli - è già stato fatto notare che si tratta di una comunità

e motore per il passaggio di un Comune da una Regione all'altra, indipendentemente dal fatto che si tratti di Regioni autonome o ordinarie,

un percorso denso di importanti punti interrogativi. Mi spiego meglio. Noi stiamo parlando qui di confini interni, ma se il criterio è questo e se la Repubblica lo fa proprio, è difficile non sostenere - anzi, a maggior ragione - che l'unitarietà dell'etnia e della nazione non deve ispirare anche la definizione dei confini internazionali. E questo criterio contrasta con tutti i motivi ispiratori dell'intera storia repubblicana nella definizione dei confini. Il Trattato fra l'Italia e l'Austria per la soluzione della questione altoatesina è fondato sul presupposto opposto; il Trattato di Osimo, che lascia di là dal confine, nella Jugoslavia di allora, nella Slovenia e nella Croazia di oggi, comunità italiane, è fondato sul presupposto opposto, ed è un presupposto contrario anche a quello in base al quale nella nostra Regione Friuli-Venezia Giulia ci sono comunità slovene e comunità nazionali nazionali tedesche, austriache. Se la Repubblica fa proprio questo criterio apre una strada pericolosa, che io credo non dobbiamo percorrere. Concludo dicendo che, sulla base di quel ragionamento, in Friuli-Venezia Giulia noi potremmo sì accogliere nel nostro territorio il Comune di Sappada, ma dovremmo dare Tarvis e Pontafel all'Austria, che noi oggi chiamiamo Tarvisio e Pontebba. E dovremmo dare - non restituire - alla Slovenia un Comune

dovremmo chiedere la restituzione di Capodistria, che in Slovenia oggi viene chiamata Koper, e la restituzione anche della croata Pola, che i croati chiamano Pula. Pula. Sulla base di questi ragionamenti, sollecito nuovamente il Governo ad adoperarsi affinché il provvedimento venga ritirato. Nel far questo, esprimo anche un giudizio politico, che non è fondato soltanto su un approccio localistico e regionalistico, ma tiene conto di come è l'Italia oggi nel contesto europeo e di quali siano le relazioni, fortunatamente molto positive e collaborative, con Stati nazionali confinanti, nei quali ci sono anche cittadini austriaci con nome italiano, cittadini austriaci di nazionalità slovena, e via di seguito. È un pezzo di storia che abbiamo deciso di superare, accantonando l'idea che i confini fossero o debbano essere definiti sulla base del criterio dell'omogeneità etnica o nazionale. Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, quella odierna è una giornata che non esito a definire storica, tanto per l'importanza del provvedimento che siamo chiamati ad esaminare, quanto per l'*iter*, a dir poco travagliato, che questo disegno di legge ha affrontato, rischiando di restare impantanato in Parlamento a causa, come specificherò meglio in seguito, di veti incomprensibili e poco lungimiranti strategie politiche. È quindi con grande emozione che intervengo in questa Aula, a più di un anno da quel 16 marzo del 2016, che ha visto compiersi un atto increscioso nei confronti non di chi ha presentato questo disegno di legge, ma dei sappadini stessi, che fiduciosi confidavano nell'inizio di un *iter* istituzionale che portasse loro quelle risposte che ad oggi non sono mai state date. Risposte che attendono dal lontano 2008. Risposte che volutamente avete scelto di rinviare.

«Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia». L'ho chiesto a tutti voi colleghi, ai Capigruppo, al Presidente del Senato, con il quale ci siamo incontrati anche con i referendari, facendomi tramite di quel comitato che ha portato nel luglio 2007 alla delibera del Consiglio comunale di Sappada n. 33, con la quale veniva formulata la richiesta di *referendum*. Un lavoro silenzioso ma efficace, ininterrotto, malgrado resistenze diverse anche da parte di chi ora ne cavalca la battaglia.

e la conseguente calendarizzazione nell'altro ramo del Parlamento che voglio credere non troverà altri strumentali ostacoli ostruzionistici. Un *referendum* il cui quesito recava: «Volete voi che il territorio del Comune di Sappada sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?». A questo quesito, lo ricordo, la popolazione sappadina ha risposto con un voto espresso il 9 e 10 marzo 2008: su 1.199 aventi diritto si sono recati alle urne 903 elettori, pari al 75,3 per cento,

a dimostrazione di come la popolazione abbia dato voce a quel sentire per il quale evidente è l'affinità con le comunità carsiche. Con esse infatti, da sempre, i sappadini condividono territorio, valori, destino ed anche disagi di chi vive in montagna, ai margini di una Regione, il Veneto, che non ha saputo ad oggi coglierne le difficoltà, l'isolamento, il contesto storico e geografico. Le motivazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, contenute nel documento di sintesi predisposto dal comitato di Sappada, sono la conferma che fin da tempi non sospetti i sappadini sono molto vicini ai friulani confinanti, ne condividono gli stessi modi di vita, le stesse leggi consuetudinarie, prospettive e speranze per il futuro, oltre ai legami etnici, linguistici e culturali. Forti quindi le motivazioni che hanno portato al superamento del doppio *quorum*: contiguità geografica, stessa struttura economica e sociale, vicinanza storico culturale.

Forte l'esigenza di autonomia, la stessa richiesta che ora sarà possibile esprimere per la Provincia di Belluno con il *referendum* nell'*election day* del 22 ottobre, autonomia che peraltro già avevo chiesto in sede di riforma costituzionale con un preciso emendamento, la cui sorte purtroppo a tutti è nota.

Ma questi anni di attesa, con false illusioni come quella del 16 marzo dello scorso anno, rischiano veramente di togliere fiducia nelle istituzioni, istituzioni fortemente in ritardo nel dare una risposta, nell'adempiere a doveri costituzionali. E non possono essere fatti sconti

L'emozione di quel 16 marzo, condivisa con i sappadini e spenta in un attimo, mi porta oggi ad essere cauta prima di esternare soddisfazione per un percorso che ha visto proprio in prima linea, con impegno costante, il lavoro di chi, al fianco dei referendari è sempre stato insieme a me, Flavio Tosi, segretario del Fare!, che ancora prima della sua espulsione - e tengo a sottolineare che di espulsione si è trattato - dalla Lega aveva sottoscritto e sostenuto concretamente i sappadini in questa loro scelta. Ha creduto e sostenuto fin da subito chi, attraverso un *referendum*, ha espresso la sacrosanta volontà di entrare a far parte di un'altra Regione, al contrario di chi non ha tenuto minimamente in considerazione le esigenze dei cittadini, della montagna, e cerca di ostacolare una battaglia di libertà, portata avanti nel rispetto delle posizioni di tutti,

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, questo provvedimento che propone il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto ed il suo passaggio al Friuli-Venezia Giulia, è sparito dall'ordine del giorno di questa Assemblea da marzo 2016, cioè da oltre diciotto mesi. Il suo approdo in Parlamento, lo scorso anno, aveva fatto sorgere non poche aspettative in capo ai cittadini di Sappada, che già attendevano questa pronuncia da più di nove anni, che il *referendum* che vide il 95 per cento dei cittadini di Sappada votare a favore del distacco è datato addirittura 2008. Siamo nel 2017 e non siamo ancora riusciti a dare una risposta a questa legittima richiesta. Dei 1.199 aventi diritto al voto, nel *referendum* comunale del 2008 votarono per il sì in 860 (il 95 per cento dei votanti); ci fu, nella sostanza, una manifestazione di volontà netta a favore del trasferimento amministrativo del Comune dalla Regione Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Una sostanzialmente univoca volontà dei cittadini, quindi, fuori da ogni discussione. Parlare del passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia significa, quindi, parlare di *referendum* e dell'importanza che attribuiamo, come forza politica, a questo importante strumento di democrazia diretta. Certo, colleghi, mi rendo perfettamente conto che, quando si parla di *referendum*, nasce, in seno agli appartenenti a molti partiti rappresentati in Parlamento, una certa dose di fastidio. La parola «*referendum*» così come «sovranità popolare» danno fastidio. Basti pensare al *referendum* disatteso sul finanziamento pubblico ai partiti: dava fastidio, come dava fastidio quello sull'acqua pubblica. Pensiamo al sabotaggio di Partito Democratico e maggioranza al *referendum* contro le trivelle, solo per citare i casi più noti. Certo, in questo caso parliamo di un *referendum* di minore rilevanza, che riguarda un solo Comune, anche piccolo, del Veneto; ma per il rispetto di questa manifestazione di sovranità popolare si sono espresse anche la Provincia di Belluno e quella di Udine. Si sono espressi favorevolmente al distacco anche i Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Chi altro si deve esprimere? Non vediamo, dunque, ragione per opporci. Ben sappiamo che in Parlamento ci sono forze politiche che non rispettano affatto la volontà popolare e non certo per ragioni di carattere geografico, storico, culturale, economico, religioso, politico o linguistico. Se andiamo a vedere, ciascuna di queste ragioni, al contrario, deporrebbe per una immediata adesione di Sappada al Friuli-VeneziaGiulia, piuttosto che al Veneto. Sembra piuttosto che la contrarietà manifestata da taluni, e da noi non condivisa, sia fondata sulla volontà di non creare un precedente giudicato pericoloso. Staremo a vedere nel prosieguo dei lavori. La mia conclusione, a questo punto, è prevedibile: il Movimento 5 Stelle è favorevole al riconoscimento del diritto di autodeterminazione di questa comunità. È favorevole a tutte le legittime manifestazioni di democrazia diretta ed è favorevole, *in primis*, all'istituto del *referendum*. Per questi motivi, valutiamo favorevolmente la proposta di distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e il suo conseguente passaggio alla Provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia.

un'altra. Discutiamo di questo forse perché i sappadini, nella loro storia, nella loro cultura, nelle loro tradizioni si sentono più vicini alla Provincia di Udine rispetto a quella di Belluno? Non credo sia solo questo il punto. È vero che la storia del Comune di Sappada porta a guardare verso il Friuli, almeno fino al 1835 - posso sbagliarmi nella data di qualche anno - ma non può essere solo questo il punto. La questione è ben più complessa. Sappada, questo Comune di confine con l'Est della nostra Regione, guarda a una Regione a statuto speciale.

ciò che è successo, perché c'è la volontà del popolo e la politica non può pensare di essere sempre autoreferenziale, di chiudersi nelle stanze

credo anche con dispiacere, che vuole andar via da una Regione ed essere allocato in un'altra. Vi pare una cosa da poco? Può la politica lasciar perdere? Inviterei la politica a prendere atto di quello che sta avvenendo, che oggi riguarda questo piccolo Comune, ma che riguarda già tanti altri. Per evitare quella che può diventare una slavina, una valanga, una difficoltà, bisogna che la politica corra ai ripari. In questo senso noi veneti corriamo ai ripari il 22 ottobre. Vogliamo dare un segnale molto forte di autonomia. Credo lo faranno tante altre Regioni,

Signor Presidente, come già altri colleghi, devo dire che siamo arrivati con gran soddisfazione a dare risposta positiva a un sentimento diffuso e condiviso una comunità che vuole appartenere al Friuli-Venezia Giulia e dal 2007 chiede di farlo. Ne è passato di tempo. Finalmente ci stiamo arrivando e con questo Governo, dopo tanti anni di stagnazione. Esprimo soddisfazione per la discussione in Aula del disegno di legge n. 951, «Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»,

molto articolato, che ha visto nella storia della comunità di Sappada diverse mobilitazioni di iniziativa popolare. Cito due esempi particolarmente significativi, come la raccolta di firme promossa dal parroco sappadino di allora, presso i capifamiglia a metà degli anni Sessanta, e il *referendum* consultivo del 2008, entrambi con percentuali di partecipazione molto alte e un pressoché totale favore (95 per cento nel 2008) per il passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia. Giulia. Le stesse due Amministrazioni regionali, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, l'una cedente e l'altra ricevente, si sono espresse positivamente sul passaggio, avallato peraltro dalle Province e dai 28 sindaci dei Comuni della Carnia. Non mancano, ovviamente, le motivazioni storiche che spiegano la genesi della proposta legandola al DNA dei sappadini, più affini alle comunità limitrofe della Carnia (Friuli-Venezia Giulia) rispetto al Veneto, per lingua (germanofona e friulana alla pari dei Comuni carnici di Sauris e Timau), cultura e storia. Vi si parla una lingua germanofona, un dialetto tedesco antico, simile a quello dei Comuni carnici di Sauris e Timau, entrambi situati in Carnia. È un'isola linguistica, quindi, che condivide una cultura minoritaria e tradizioni secolari con isole sorelle del Friuli. Vi convive anche la lingua minoritaria friuliana. Ricordiamo che l'annessione al bellunese è avvenuta sotto l'Impero ausburgico nel 1852, pertanto da considerarsi, a ragion veduta, recente, se si considera che il rapporto con la diocesi di Udine è stata una costante nel corso di secoli, di cui oggi fa ancora parte. da ricordare che nella Grande guerra la popolazione civile sappadina partecipò al rifornimento delle truppe sul fronte orientale con il movimento passato alla storia come quello delle «Portatrici carniche», che rischiavano la vita salendo sul fronte a foraggiare le truppe. Anche nel secondo conflitto mondiale, nel 1944, Sappada prima dell'arrivo delle truppe alleate fece parte della Repubblica libera della Carnia. Per venire ad oggi, evidenzio che i rapporti culturali ed economici di Sappada, orientati nettamente al Friuli-Venezia Giulia, sono forti e quotidiani. È da evidenziare, per quanto attiene le motivazioni più vicine a noi, che anche in ambito sportivo Sappada vive una integrazione con il Friuli-Venezia Giulia piuttosto che con il Veneto. Basti pensare che l'associazione sportiva di sci nordico Camosci, da cui sono usciti noti campioni internazionali del calibro di Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, Marina Piller, Lisa Vittozzi e molti altri, ha sempre fatto parte del comitato Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso dicasi per lo Sci Club Sappada, sodalizio di sci alpino che fa parte del comitato Friuli Venezia Giulia e, infine, della locale ASD Calcio Sappada, che da sempre milita nel campionato carnico. Anche dal punto di vista strategico e militare, Sappada è parte del Friuli. Fino a pochi anni fa vi era infatti a Sappada una caserma della Brigata Alpina Julia (non del Cadore): la caserma Fasil, ora dismessa. Infine, voglio sgombrare il campo da qualche perplessità già sollevata in sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali che riguarda un possibile effetto domino, quello prima citato dal senatore Sonego: effetto domino di richieste di passaggi da una Regione ad un'altra, investendo non tanto il provvedimento in esame quanto l'articolo 132 della Costituzione. Osservo, perciò, che l'articolo costituzionale prevede tanti e specifici presupposti per il distacco-aggregazione di un ente locale da rendere improbabile che la sua applicazione diventi generalizzata. Infine, su tutte queste premesse e considerazioni ritengo non ci siano ragioni ostative al passaggio del Comune di Sappada, della comunità di Sappada,

che, soprattutto, debba essere rispettata da più parti richiamata volontà dei cittadini, che sono stati molto chiari e decisi, e per molti anni, nella loro intenzione di voto. Cittadini le cui aspettative non possono essere deluse. Misure di cautela e di procedura hanno determinato in passato un rinvio,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò dei fatti di Bagheria. Il 7 e l'8 aprile del 2015 il sindaco di Bagheria, attivista del Movimento 5 Stelle, già stretto collaboratore di Giancarlo Cancelleri, deputato all'Assemblea regionale siciliana ed oggi candidato a Presidente, affida alla Tech Servizi Srl la gestione straordinaria del servizio di raccolta di rifiuti per il Comune di Bagheria. Solo che lo fa senza gara e per sei mesi, per un importo di 500.000 euro più IVA al mese: troppo e troppo a lungo. Parte dell'opposizione in Consiglio comunale ha fatto una dura battaglia contro questi provvedimenti, chiedendo l'intervento degli assessorati regionali competenti che, in effetti, il 15 aprile successivo mandano una nota nella quale si evidenzia la dubbia regolarità del procedimento. L'amministrazione comunale di Bagheria procede comunque senza tentennamenti sulla strada decisa, mentre la Regione siciliana, nonostante le segnalazioni anche formali delle opposizioni, non si attiva efficacemente. In effetti, il Movimento 5 Stelle nella attuale legislatura regionale siciliana è stato spesso accusato di collateralismo con l'amministrazione Crocetta. Fatto sta che la Regione ha mostrato un torpore profondo verso le modalità di gestione del Comune di Bagheria da parte del Movimento 5 Stelle, nonostante le reiterate segnalazioni delle opposizioni. Il 24 settembre 2015 viene presentata una interrogazione a mia prima firma, rivolta al Governo per sapere se tali fatti sono noti e, se sì, cosa si intenda fare. Tale interrogazione è stata più volte sollecitata, fino ad oggi inutilmente. Io stesso, allora, presento un esposto ai carabinieri di Bagheria il 2 novembre 2015. Di oggi è la notizia di una serie di provvedimenti della magistratura che hanno raggiunto il sindaco di Bagheria e alcuni assessori e funzionari del Comune. Da questi fatti traggo due considerazioni, che vi sottopongo. La prima è che il Movimento 5 Stelle deve riconsiderare il proprio atteggiamento nella gestione concreta della cosa pubblica, se vuole essere credibile come forza di governo, anche nel rapporto con le opposizioni. La seconda è che tutta la politica ha bisogno di riprendere a funzionare correttamente: i ritardi da parte di chi doveva operare i controlli amministrativi (la Regione) e da parte degli organi periferici dello Stato e i ritardi del Governo, che ad oggi non ha risposto, hanno lasciato un'enorme responsabilità di supplenza alla magistratura. Il controllo della politica deve avere maglie assai più strette rispetto a quelle penali. La tempestiva e puntuale condanna politica di certi atteggiamenti amministrativi

Signor Presidente, sono passati pochissimi giorni dalla drammatica morte di Noemi Durini, la ragazza di Specchia che è stata barbaramente uccisa. Oggi ci troviamo, ancora una volta, davanti a un altro tragico episodio, che ha ridotto una giovane donna in fin di vita, veramente in condizioni disperate. Si tratta di una ragazza di quindici anni di Ischitella, in provincia di Foggia, ferita brutalmente da un uomo che poi si è suicidato: ferita da un colpo di pistola in pieno volto. Parliamo quindi di un altro episodio che apre uno scenario veramente macabro di violenza e di paura. evidente che ci troviamo davanti a un allarme veramente importante, che deve trovare i giusti strumenti per essere finalmente placato. Non possiamo assolutamente continuare a piangere vittime e abusi continui. Quante altre morti serviranno per prendere atto di questa situazione e di questa emergenza, perché ormai si tratta di una vera e propria emergenza? Quante altre volte, quanti altri giorni, mesi, anni dobbiamo aspettare perché questo Governo intervenga finalmente, facendo delle buone azioni, tutelando il territorio, aiutando i cittadini? Stiamo parlando di stragi senza arresto, che giorno dopo giorno hanno assunto una portata veramente spaventosa. La violenza di genere infatti rappresenta la prima causa di morte tra le donne. Il Governo dov'è, mentre si compie questo massacro? Perché le reti territoriali non vengono rafforzate e messe nella condizione di lavorare in sinergia con le altre? Perché non c'è una lungimirante programmazione degli interventi e lo stanziamento di adeguati fondi e risorse? Domande a cui segue un silenzio imbarazzante, perché l'Esecutivo è assente. Non dimentichiamo che lo scorso luglio è scaduto il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e il fatto che le istituzioni temporeggino sull'argomento è a dir poco scandaloso. Ormai anche uscire dalla porta di casa per andare a scuola, per fare acquisti, per fare semplicemente una passeggiata significa esporsi a un pericolo concreto per la propria incolumità. Tutto questo è davvero inaudito per una società che si definisce evoluta. Non c'è più tempo, non si può aspettare ancora, non si può indugiare su un tema così delicato. Una cosa è certa: in questa situazione ogni altra vittima ricadrà sulla responsabilità dello Stato e di chi non interviene, cioè voi.

In quest'interrogazione chiedo una risposta urgente del Ministero, perché il 13 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione ha emanato i requisiti *standard* e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specialità dell'area sanitaria, in particolare stabiliti dall'Osservatorio nazionale di specializzazione medica. Questi *standard* specifici appaiono assolutamente incongrui alle realtà cliniche presenti e ciò ha fatto sì che molte scuole hanno dovuto inserire dati esageratamente ottimistici o entusiastici per poter essere all'interno di tali *standard* e quindi avere la possibilità di formare

ottima offerta formativa che si trovano ad avere ottemperato ai requisiti richiesti dal Ministero, ma che non potranno avere un numero di studenti così come negli altri anni era successo. Sollecito quindi la risposta perché, dovendo in

Non entro nei dettagli per ragioni di tempo, ma vorrei sottolineare che la presidente della Federazione degli ordini dei medici, Roberta Chersevani, ha proposto ieri di spostare le guardie mediche all'interno delle stazioni dei carabinieri o nei commissariati di polizia

via. Si tratta di un problema che va sicuramente affrontato e approfondito, come ha chiesto in questi giorni la presidente Boldrini, che ha esortato le forze politiche a mettere in campo un provvedimento in cui si aumentino le tutele a favore delle donne e le misure interdittive per gli uomini violenti. È un dovere e una responsabilità alla quale la classe politica non può e non deve sottrarsi. **Per